L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

accadimenti che si stanno sviluppando in queste ore praticamente in tutta la nostra Penisola, connessi con l'ondata di maltempo che sta abbattendosi su diverse parti del nostro Paese con delle ripercussioni molto pesanti. Le cronache di questi minuti ci riportano situazioni drammatiche in Sicilia, con l'intera città di Catania al buio senza l'erogazione di servizi

la drammatica situazione della Lombardia; anche questa notte Milano è stata colpita da trombe d'aria. Purtroppo una ragazza di sedici anni in Lombardia ha perso la vita a seguito del crollo di un tronco d'albero. Milano, l'*hinterland* milanese, la città metropolitana e la Brianza sono state pesantemente colpite con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini, sull'erogazione dei servizi e sulla mobilità. Anche in Emilia-Romagna, purtroppo nelle zone alluvionate, si sono riscontrati fenomeni di questa natura. Nel Veneto abbiamo una pesante situazione che ha coinvolto purtroppo un ragazzo di sedici anni, ferito gravemente. gravemente. Il cambiamento climatico si impone e i fatti sono evidenti e sempre più sotto gli occhi di chi li vuole vedere. Riteniamo indispensabile - mi rivolgo al Governo che è presente

Manifestiamo, naturalmente, la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a tutte le popolazioni colpite e alle famiglie che devono purtroppo contare e piangere i propri morti e chiediamo anche una particolare attenzione e sensibilità da parte del Governo affinché lo stato di emergenza che, come abbiamo visto, verrà richiesto da parte di diverse Regioni, venga rapidamente deliberato per venire incontro alle problematiche specifiche. Dopodiché, c'è un tema più generale, che naturalmente rimanda alla questione di una legge sul clima che non può più essere rinviata.

colpire le fasce più deboli delle nostre popolazioni.

colpite e rivolgere un pensiero di profonda gratitudine a tutti coloro che si sono attivati nei soccorsi sul posto che, come sempre, vedono all'opera le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco

il Governo in tutte le attività che potranno rendersi necessarie, nel decretare lo stato di emergenza ove questo sia necessario e opportuno.

una gestione dell'acqua che è stata troppo trascurata nel passato, con tutte le conseguenze che vediamo, mettendo in campo i famosi laminatoi e tutti gli strumenti che possono servire da un lato a combattere la siccità, di cui parlavamo fino a poche settimane fa,

anche noi ci uniamo alla richiesta di una informativa urgente del ministro Musumeci. Questa notte in provincia di Brescia - la mia Provincia - una ragazza di sedici anni ha perso la vita travolta da un albero per un forte temporale mentre era in un campo *scout* in Val Camonica. Ieri una donna è morta per un albero caduto in provincia di Milano. Questa notte

di una serie di episodi di maltempo che stanno affliggendo l'Italia e che non si sono mai registrati con questa intensità negli ultimi dieci anni, come dice lo stesso ministro Musumeci. L'Italia è spaccata in due: ci sono incendi in Sicilia, sappiamo che gli aeroporti di Palermo e di Catania sono chiusi; la città di Catania è alle prese con difficoltà di distribuzione dell'acqua potabile, perché non c'è l'energia elettrica a causa del grande caldo; a Palermo sappiamo che una donna è morta perché gli incendi hanno impedito ai soccorritori di andare a soccorrerla a casa sua, dove aveva avuto un malore; un malore; al Nord Italia la circolazione ferroviaria è interrotta per il maltempo; la Lombardia ha chiesto lo stato di calamità naturale; la Coldiretti ha chiesto anch'essa lo stato di calamità naturale, perché le coltivazioni in Lombardia sono state distrutte dal maltempo. Io credo che la fenomenologia di queste ore e di questi giorni ci dimostri dobbiamo fare i conti con un cambiamento climatico che sta modificando le nostre vite. Oggi dobbiamo fare i conti con l'emergenza e chiediamo al ministro Musumeci di venire a riferire in Parlamento, ma credo che la politica tutta debba interrogarsi su come gestire questo cambiamento climatico, che rischia di cambiare le nostre vite in maniera drammatica. Chiediamo adesso che il Ministro venga a riferire, perché questi sono episodi allarmanti e drammatici e, nel fare questa richiesta, ovviamente ci stringiamo con affetto ai familiari e ai parenti delle vittime di questo straordinario episodio di maltempo.

ho fatto fatica a fare il giro della casa per chiudere tutte le finestre, perché stava accadendo qualcosa che io non avevo mai visto in vita mia e non ho dodici una violenza incredibile, uno scroscio d'acqua associato a un vento fortissimo. La sensazione era proprio quella della violenza straordinaria, mai vista prima. Non ho potuto far altro che far correre pensiero a quest'Aula e alle discussioni che si stanno facendo. Mi rendo conto che forse è difficile cambiare la versione e la propria prospettiva; proviamo a cambiare nome se vi dà fastidio l'espressione cambiamenti climatici, ma non si può fare a meno di constatare quello che di fatto avviene. Chiamatele come volete, ma non sono cose

che sono un patrimonio perso per sempre, che non si riesce a ricostruire in una città densa di cemento e che non riesce più ad accogliere questi alberi. La prospettiva futura che abbiamo è veramente seria e grave. Pertanto, se non vogliamo chiamarli cambiamenti climatici,

competenze scientifiche per lavorare sulla prevenzione in modo adeguato: bisogna conoscere il territorio e le ripercussioni delle attività antropiche sul territorio collegate a questi eventi straordinari. Sto pensando alle infrastrutture costruite in luoghi non idonei, che hai voglia di ricostruirle, ma, se dopo due mesi si ripete lo stesso episodio, avremo lo stesso risultato. Quindi il ragionamento della prevenzione dobbiamo farlo con i tecnici, perché possano valutare le situazioni di pericolosità del territorio e capire come agire. L'unica via che abbiamo è la prevenzione, ma per farla occorre fare investimenti ed entrare nell'ottica che questa è la priorità.

calamitosi incredibili, che non avevamo mai visto, e ripetuti; la cosa che ci preoccupa di più è questo. Tanto è vero che molti colleghi mancano oggi proprio perché non sono riusciti ad arrivare. Quindi un abbraccio va sicuramente alle popolazioni colpite, dalla Lombardia all'Emilia-Romagna, al Veneto e alla Sicilia, che ha invece il problema degli incendi. Vogliamo dire un grazie innanzitutto alla gente e alla popolazione, perché quando sono tornata a casa i tetti erano già coperti con i teloni di nylon. Ma ci hanno chiesto aiuto immediato, loro e i sindaci. I sindaci sono delle persone che devono fare da aiuto psicologico a quelle persone, che si trovano senza niente. Serve sicuramente un intervento del Governo, in aiuto dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Ci sono tanti immobili comunali danneggiati, quindi sicuramente il Ministro e la stessa presidente Meloni faranno un intervento che stia a dimostrare la vicinanza di questo Governo, anche in un momento così difficile per il nostro Paese.

ho assistito direttamente, venerdì sera a Brugherio e ieri mentre stavo andando a Milano, al cambiamento radicale che è avvenuto. Però questo è un dato;

non le ho mai viste con tanta violenza e con tanta rapidità di cambiamento. È necessario affrontare questo tema. È chiaro che è necessario essere vicini alle popolazioni ed è necessario stanziare immediatamente risorse per affrontare tali questioni. Il dato è anche un altro: molto spesso i Comuni si trovano da soli ad affrontare questo tema e non hanno le risorse sufficienti

Grazie, queste emergenze, una volta che si ripetono con continuità, non sono più emergenze e che richiedono interventi strutturali, una programmazione di cose da fare. Questo ragionamento mi pare molto lontano soprattutto dall'opinione di diverse persone che in parte siedono in quest'Aula e che ancora non si sono convinte che ci muoviamo verso una direzione da cui non sarà più possibile tornare indietro. Colleghi, quando un Ministro tedesco l'idea che magari un domani bisognerà andare a fare turismo nel Mare del Nord perché nei mari del Sud farà troppo caldo, è inutile arrabbiarsi. Bisogna fare fronte alla situazione e prepararsi a estati in cui farà più caldo; prepararsi significa avere le infrastrutture, avere l'acqua, avere la possibilità di offrire un soggiorno adeguatamente piacevole a quelli che dovessero scegliere il nostro Paese. sia possibile, bisogna evidentemente intervenire in modo strutturale con un piano che francamente non ho ancora visto.

il cordoglio e la vicinanza alle popolazioni colpite. Il ringraziamento va anche alle forze che sono già intervenute. Contattata informalmente la segreteria del ministro Musumeci, ci ha dato la disponibilità, non appena possibile, a venire a riferire e credo che vi sarà un contatto con la Presidenza in questo senso. Ricordo fra l'altro che domani, alle ore 19, è previsto un Consiglio dei ministri e quindi una valutazione, anche alla luce della ricognizione, potrà essere più articolata e immediatamente affrontata da parte del Governo.

c'è stato un incontro anche con l'Intergruppo parlamentare su Expo 2030. In quell'occasione, insieme al collega Verini (entrambi facciamo parte dell'Intergruppo), è nata l'idea di presentare una mozione affinché il Parlamento Parlamento possa sostenere la candidatura di Roma per Expo 2030. Voglio quindi ringraziare tutte le forze politiche, nessuna esclusa, tutti i Gruppi presenti in Senato hanno sottoscritto tale mozione e credo che questo sia un fatto molto importante. Voglio anche segnalare che il punto 3 della mozione deve essere soppresso, in quanto sostanzialmente un tavolo permanente già esiste, quindi di fatto oggi quel punto è superato. Resta l'importanza di questa mozione nel sostenere una candidatura che riteniamo strategica, che nasce nel 2020. Voglio qui ricordare che, insieme all'assemblea capitolina, vale a dire il consiglio comunale della capitale, proprio Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio attuale, allora consigliera capitolina,

voglio ricordare che in occasione delle elezioni amministrative del 2021 tutti i candidati sindaci di ogni parte politica avevano inserito nel programma il sostegno a Expo 2030,

per la capitale: penso alle Vele di Calatrava, un'opera interrotta nata in teoria per i mondiali di nuoto del 2009 e rimasta a rappresentare invece tutt'altro. Si tiene conto della grande potenzialità dell'opera dal punto di vista sociale, economico ed ambientale per l'area individuata, un'area

rappresentare una localizzazione ideale, anche perché ha adeguati spazi e adeguate potenzialità anche dal punto di vista del trasporto pubblico e dei servizi da da realizzare. Si tratta, tra l'altro, di un'area nella quale si può immaginare, anche dal punto di vista ambientale, uno straordinario corridoio che dal Parco del Colosseo, dal Palatino, passando per il Parco dell'Appia antica e per quello degli acquedotti, arrivi fino all'area

ma che va giocata fino in fondo. Da questo punto di vista voglio anche ringraziare, perché so che è sensibile su questo, il presidente dell'UIP, senatore Casini, perché è importante che anche chi tra noi ricopre ruoli internazionali li sappia giocare fino a novembre, che è il

la cultura, l'arte, l'enogastronomia, la moda, tutto ciò che rende l'Italia unica nel mondo. Abbiamo il sogno che è stato rappresentato da Roma nei secoli a livello universale. Ora sta a noi impegnarci fino all'ultimo minuto, affinché quel sogno possa divenire la realtà della sfida di Expo 2030 assegnata a Roma e all'Italia. *(Applausi)*. come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 18 luglio, per tutte le mozioni all'ordine del giorno la discussione sarà limitata alle sole dichiarazioni di voto, per un tempo di cinque minuti a Gruppo.

così importante come Expo 2030. Siamo davvero molto compiaciuti per i consensi che la città di Roma sta ottenendo, caro senatore De Priamo. De Priamo. Personalmente, sono impegnata proprio direttamente in una serie di bilaterali a supporto dell'azione del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri. anche sottolineare come non sia solo un impegno circoscritto, perché viene invece portato avanti davvero da tutti i Ministeri, ciascuno per la propria tematica. È stato già detto molto e bene da parte del senatore De Priamo, però credo in aggiunta dobbiamo essere tutti consapevoli che è davvero un appuntamento imprescindibile per la nostra Capitale.

mi pregio di informare anche gli onorevoli senatori che ci sono state alcune iniziative mirate *ad hoc* in tutte le manifestazioni internazionali

Vi ringrazio e speriamo davvero di rimettere la nostra straordinaria Capitale al centro di tutte le iniziative di questa caratura.

quella presente è un'occasione straordinaria, probabilmente irripetibile, anche perché, se legata magari anche all'evento giubilare che ci sarà nel 2025,

un'esposizione internazionale e mondiale come l'Expo in termini di capacità d'ingresso nella nostra società di visitatori e di introiti in positivo dal punto di vista economico (parliamo infatti della possibilità d'ingresso di circa 50 miliardi,

un'unità di intenti non solamente per Roma, ma per tutta l'Italia. È per questo motivo che il nostro Gruppo voterà a favore e a sostegno della mozione.

che questa mozione sia stata sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari e che ci sia quindi un impegno comune di tutto il Parlamento per sostenere la candidatura di Roma all'Expo 2030. Naturalmente, penso di potermi associare a quello che è stato detto: è effettivamente un'opportunità

Signor Presidente, anche noi ovviamente siamo a favore di questa mozione, perché - come è già stato detto - è un'opportunità straordinaria per il nostro Paese, oltre che ovviamente per la città di Roma. L'Expo non è soltanto da considerarsi una vetrina per quanto di buono siamo in grado di produrre in Italia, ma è anche e soprattutto un'opportunità di riflessione interna sul miglioramento del nostro modo di gestire la città e il nostro Paese. È come quando si invita a casa un ospite importante: gli si fa trovare la casa in ordine, il bagno pulito, gli si trovare gli elettrodomestici che funzionano e la stanza degli ospiti perfettamente adatta ad ospitarlo. Ecco, questo dovrebbe avvenire anche per noi, anche per Roma. mi auguro che si colga una tale occasione per la nostra città di adozione - non siamo romani, ma siamo qui a svolgere una funzione a cui ci ha delegato il popolo italiano italiano - per rimettere in gioco alcuni suoi meccanismi di funzionamento e per presentarsi all'altezza della situazione. Avremo visitatori da tutto il mondo, avremo la possibilità di far vedere che abbiamo non solo sassi e monumenti, ma anche la capacità di tenerli in modo adeguato ai tempi e a coloro che ci visiteranno. Signor Presidente, non mancheremo di far avere il nostro sostegno alla candidatura di Roma per Expo 2030 e ringrazio la sottosegretaria Tripodi, per aver pronunciato parole importanti importanti di impegno del Governo su tale candidatura, che ovviamente è sostenuta da tutte le forze parlamentari, come è giusto che si faccia quando è l'Italia ad essere in gioco. Non si tratta solamente di un'occasione storica per la Capitale del nostro Paese: è un'occasione storica per il nostro stesso Paese, intanto perché la candidatura si lega a un altro evento importante come quello del Giubileo del 2025 e poi perché - come ricordato dai colleghi -l'indotto che verrà prodotto, con quasi 300.000 posti di lavoro, 50 miliardi di euro, equivalenti a 3 o 4 punti percentuali di PIL, avrà un effetto importante non solo sul turismo, ma anche sull'intera nostra economia e sul nostro territorio. Proprio perché vogliamo arrivare preparati a questo appuntamento di novembre, sono molto d'accordo con le parole prima esplicitate dal senatore Spagnolli, oltre al lato degli investimenti e della promozione, la cosa più straordinaria che questa città deve imparare a fare è avere cura della propria bellezza. E la cura della propria bellezza la si pratica quotidianamente, attraverso l'amministrazione, attraverso la raccolta differenziata, attraverso la pulizia nei centri storici e nelle aree degradate e più periferiche, attraverso l'inclusione, attraverso l'accessibilità. È vero che dobbiamo essere unitari quando, a livello internazionale, sosteniamo la candidatura, ma questo non ci può esimere anche dall'essere molto netti quando affrontiamo i problemi di una città nella quale ormai prendere un taxi è diventata un'impresa, in cui trovare un luogo nel quale

di sostenere la candidatura a Expo 2030. Altrimenti, il passaggio dall'essere commissari all'essere commissariati rischia di essere davvero breve. Quindi, sì al sostegno unanime alla mozione sulla candidatura di Roma, ma anche la richiesta di un impegno quotidiano, perché abbiamo ricevuto le bellezze di questa città in eredità ma dobbiamo ancora dimostrare di esserne in grado.

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il Gruppo Forza Italia sostiene con convinzione questa mozione, che io stesso ho sottoscritto come parlamentare l'altro, di essere quello con il mandato più lungo e longevo nell'ambito della Capitale. Noi riteniamo che l'occasione dell'Expo 2030 debba essere colta dalla Capitale. questo atto del Parlamento, che con il collega De Priamo e altri colleghi abbiamo voluto e sostenuto, è un momento di sostegno ulteriore all'azione che il Governo sta profondendo. Anzi, proprio in questa occasione devo sottolineare l'azione dell'intero Esecutivo e anche l'incisiva azione del ministro degli esteri e vice presidente del Consiglio, Consiglio, Tajani. Peraltro, qui oggi abbiamo il sottosegretario Tripodi che rappresenta il Governo e il Ministero degli esteri in particolare. L'azione del presidente Tajani, d'accordo con il presidente del Consiglio Meloni, che pure sta agendo personalmente e direttamente per questo obiettivo, ha attivato tutta la nostra rete diplomatica, le ambasciate, i consolati, le camere di commercio e tutte le realtà degli italiani all'estero per una campagna che possa portare alla assegnazione della Expo a Roma. Le ragioni non dobbiamo particolarmente illustrarle, nel Parlamento italiano e nel Senato della Repubblica ospitato nella città di Roma. La Capitale, con il Giubileo e con altri eventi, è già al centro del protagonismo internazionale. Le potenzialità, sotto il profilo dell'accoglienza, sotto il profilo del risalto che l'Expo potrebbe avere sono enormi.

nell'agenda delle opere pubbliche, anche del PNRR e degli obiettivi che le amministrazioni locali, ma anche lo Stato, devono realizzare. Tra l'altro, noi stiamo anche discutendo, sperando che questa sia la legislatura giusta, di dotare la Capitale di poteri specifici,

concepiamo la mozione in esame come un momento di sostegno alla campagna e alle iniziative che il Governo sta promuovendo, come con l'azione della *task force*. Sappiamo che ci sono altri concorrenti importanti. Comprendiamo perfettamente le aspirazioni della città di Odessa

Siamo reduci dalle vicende qatarine in Europa. Ci auguriamo che la competizione su questa vicenda sia leale e trasparente tra Stati e progetti, perché la ricchezza di alcuni luoghi è frutto delle materie prime e delle risorse che essi hanno. Spesso ne abbiamo visto emergere quantità notevoli e abbiamo visto anche tanti eventi sportivi e non sportivi camminare là dove la ricchezza li richiama. Questo accade nella storia dell'umanità e non ci scandalizziamo. Quindi, rispettiamo tutti i concorrenti di Roma. Non poniamo la candidatura di Roma su un piano di storia millenaria e plurimillenaria, perché anche altri luoghi del mondo hanno le loro storie e le loro tradizioni, che noi rispettiamo. Ci auguriamo però che il voto convergente e unanime del Senato e del Parlamento dia ulteriore forza all'azione del Governo in attesa dei momenti decisivi e delle procedure che dall'autunno daranno luogo alle decisioni. Forza Italia

Signor Presidente, sottosegretaria Tripodi, anche io come parlamentare romana ho immediatamente sottoscritto e sostenuto l'idea di questa mozione per dare maggior vigore all'impegno del Governo e di tutti gli enti e gli organismi che hanno potere di farsi ambasciatori

ha attraversato diversi Governi e diverse amministrazioni locali. Credo che anche questa mozione, sostenuta in maniera trasversale da tutte le forze politiche, sia la dimostrazione del fatto che si prova, per una buona causa, a unire le forze affinché la candidatura di Roma possa a novembre - una scadenza ormai prossima - andare a buon fine. Come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, la competizione è aspra, la competizione è aspra, può essere anche scivolosa, ma la candidatura di Roma ha moltissimi punti di forza dalla sua. Non starò a ripetere quanto è ovvio, cioè la cultura e la bellezza che caratterizzano la nostra Capitale dall'alba dei tempi.

i padiglioni che poi, anche una volta cessata la manifestazione, possono essere con pochi ritocchi ritrasformati e quindi essere utilizzabili per il territorio, in parte dalla stessa università, dal policlinico. Si tratta un Expo a impatto zero perché si mira ad avere una manifestazione e una *location* che siano del tutto autonome dal punto di vista energetico, senza ulteriore impatto

che da Roma si dirameranno poi all'intero Paese; si stimano circa 300.000 posti di lavoro e probabilmente proventi

tra i 179 Paesi che poi dovranno alla fine votare. Annuncio con questo il voto favorevole del mio Gruppo MoVimento 5 Stelle Signor Presidente, anche noi abbiamo sostenuto e promosso questa iniziativa. Facciamo parte dell'intergruppo parlamentare di sostegno a questo obiettivo che rappresenta una vera e propria sfida

mozione. Non voglio ripetere cose che condivido: è una grande occasione non solo per Roma, per l'Italia centrale, ma per il Paese intero, come si dice per il sistema Paese. Paese. Ci sono investimenti di miliardi, ci sono posti di lavoro e ci sono occasioni di innovazione: è quindi una sfida a

occasione - anche quella - di dialogo. Sappiamo come qui a Roma le religioni monoteiste si sono incontrate da sempre e il Giubileo sarà un'altra occasione per

un ruolo davvero importante per poter aiutare i Paesi del mondo, come sta avvenendo nelle ultime ore con il convegno alla FAO sugli obiettivi Fame zero 2030. Ancora una volta Roma guarda al futuro e non soltanto al proprio passato. Ancora una volta questa Capitale dà un contributo non provinciale ma davvero globale. Non sappiamo se il progetto

Signor Presidente, colleghi, Roma è da sempre lo specchio e la vetrina del Paese; ogni anno è meta di milioni di turisti che da ogni parte del mondo giungono alla scoperta delle testimonianze della città che può a buon diritto considerarsi la culla della civiltà occidentale. Roma è anche il centro del Cristianesimo, il luogo dove la fede in Cristo si è istituzionalizzata e ha costruito intorno alla Chiesa un patrimonio unico di cultura, valori e testimonianze artistiche. Per queste ragioni, Roma, che non a torto è stata chiamata la città eterna, non può essere abbandonata a sé stessa, non può soccombere alla devastazione e al degrado che sono l'ineluttabile destino cui la condannano il disinteresse e l'incuria in cui è stata lasciata per troppi anni. Il riscatto di Roma è nelle nostre mani, nelle mani - intendo - della politica e del buon governo, nella nostra capacità di fare scelte coraggiose e lungimiranti. L'occasione che Roma sia designata come la città ospitante l'Esposizione universale del 2030 è perciò assolutamente da non perdere. L'Expo può rappresentare lo stimolo migliore per generare - come è avvenuto a Milano - un circolo virtuoso in cui tutti facciano la loro parte per il riscatto della città: le istituzioni pubbliche, i privati, il mondo dell'industria e delle professioni, i comuni cittadini. I dettagli dell'effetto a catena che l'evento potrebbe generare sono illustrati con chiarezza nella mozione; in questa sede mi limito a dire che l'Expo ci permetterebbe di ridisegnare finalmente la città, di porre mano ai necessari interventi strutturali e infrastrutturali di cui ha bisogno. Non dimentichiamo, però, che il problema di Roma e dell'Italia è anche e soprattutto culturale. Negli ultimi anni ha trionfato una cultura del no che ha immobilizzato le nostre energie, che ci ha tarpato le ali. Occorre adesso una cultura del fare, del progetto, del buon senso e della concretezza. E questo per noi della Lega è un dovere primario, la risposta migliore a chi vuole rinchiuderci nei recinti asfittici di una decrescita che non sarebbe affatto felice. A Roma, in particolare, ci si è spesso trincerati dietro l'alibi di un patrimonio storico e archeologico da tutelare, quasi che non fossero gli interventi umani ad aiutarne la conservazione e a promuoverne la valorizzazione. Solo in un rapporto vivo con il presente, il passato può continuare a esserci da esempio. La storia stessa di Roma ci dice, d'altronde, che la città si è conquistata la fama di essere eterna proprio grazie alla capacità, che ha dimostrato in certi momenti, di sapersi rinnovare in uno spirito di continuità, ma anche con la capacità di ragionare in grande. Penso all'età barocca, quando i geni artistici di Bernini e Borromini dettero alla città nuova linfa e vigore e ne rinnovarono le antiche glorie. la possibilità che ci dà l'Expo è troppo importante per il nostro Paese per concederci distrazioni. Con la mozione n. 54 vogliamo impegnare il Governo tutto e impegnarci noi in prima istanza affinché, con le opportune azioni nei luoghi deputati, la candidatura di Roma vada in porto. Mostriamo per una volta tutti insieme di essere coesi su un obiettivo di puro interesse nazionale, perché la reputazione internazionale del Paese e la rinascita dell'Italia passano anche attraverso il rilancio economico, culturale e sociale di Roma. Per tutto questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega.

essere un rilancio notevole e rilevante per la cittadinanza italiana. Si tratta di una grande occasione per Roma, che si andrebbe a stagliare immediatamente dopo il grande Giubileo del 2025, sul quale tanto impegno stanno approfondendo la città e il Governo. Noi auspichiamo fortemente che questa possa essere anche una grande occasione per la Capitale, che sicuramente ha bisogno

e per questo, ad esempio, io vorrei richiamare il primo provvedimento importante per la città di Roma che è derivato dal finanziamento di un infrastruttura trasportistica rilevantissima. Non sfuggirà che, per avere la possibilità di anelare a essere prescelti in contesti internazionali di tal genere, è bene che Roma si faccia trovare pronta. È per questo che il Governo Meloni scelse di finanziare, in un bilancio scritto per dieci dodicesimi da chi ci ha preceduto, la metro C, che è la grande infrastruttura trasportistica che deve collegare il Sud e il Nord della città, per rendere Roma adeguata a quelle che sono le altre grandi capitali europee.

l'Expo 2030. Penso ai 30 milioni di visitatori che arriveranno in Italia, che sicuramente porteranno ricchezza e crescita a livello nazionale. Penso alle 11.000 aziende che potranno operare e lavorare, alle grandi infrastrutture che vi ruoteranno intorno, ai 300.000 posti di lavoro che si potranno andare a creare.

È il fatto che credo che nessuna città al mondo sia in grado di accogliere la grande esposizione volta allo sviluppo delle scienze e delle tecnologie umane come può essere accogliente Roma, la nostra Roma, con quello stratificarsi straordinario di storia, di cultura e di arte che l'ha resa nota nel mondo come la città eterna, che ha un filo conduttore che ha sempre unito i secoli agli altri, quella tradizione eccezionale

Poiché ci sono colleghi ancora impegnati nella seduta della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, non procediamo al voto,

un elemento di grande preoccupazione attorno a questo disegno di legge sull'autonomia differenziata. Il Ministro lo sa bene; ne abbiamo discusso molte volte nel corso delle ultime settimane. La preoccupazione - se posso riassumerla in una battuta, anche per i tempi molto stretti di questa illustrazione - è che in un Paese come il nostro, già profondamente segnato dal divario territoriale e dalla diseguaglianza - elementi che peraltro dopo la pandemia sono cresciuti in maniera esponenziale e che caratterizzano da molti decenni la vita dell'Italia - questo disegno di legge del ministro Calderoli sull'autonomia differenziata possa accentuare in maniera molto profonda questi elementi di divario territoriale. E quindi, invece di favorire quella coesione territoriale che oggi servirebbe per mettere il Paese nella condizione di essere maggiormente competitivo su scala europea, temiamo possa aggravare una situazione che evidentemente è già molto compromessa. Lo dico semplicemente per spiegare di cosa parliamo quando trattiamo dei divari territoriali. Parliamo di un Paese in cui, signor già tra il Nord Italia e il Sud Italia addirittura l'aspettativa di vita delle persone non è la stessa: l'aspettativa di vita di un cittadino meridionale è di quattro anni inferiore a quella di un cittadino Capite bene che, dinanzi a una situazione così clamorosa, che naturalmente si è accumulata nel corso degli anni se non addirittura dei decenni, oggi avremmo l'assoluta necessità di provare a capire di provare a capire quali elementi potrebbero essere funzionali a mettere in discussione questi dati strutturali e a determinare una qualche inversione di tendenza. La forte preoccupazione, in particolare delle forze politiche di opposizione - tra l'altro, questa mozione è firmata non semplicemente da me, ma da tre Gruppi parlamentari e questo mi sembra mi sembra un fatto politico molto significativo - è che questi elementi di maggiore diseguaglianza e di maggiore divario possano essere accentuati se il disegno legge Calderoli dovesse effettivamente arrivare a compimento così come è iniziato. Ovviamente, è inutile dire che spero e mi auguro che già oggi, discutendo questa mozione e interloquendo con il Governo, ma anche quando passeremo al voto degli emendamenti, almeno alcuni degli emendamenti dell'opposizione possano essere effettivamente presi in considerazione e si possa cercare di dare un altro segno al provvedimento. Vorrei dire anche che, che, per quanto questo disegno di legge è dal mio punto di vista particolarmente critico per il Mezzogiorno del Paese, penso vada guardato anche con un elemento di preoccupazione non semplicemente per il Sud. Credo infatti che l'autonomia differenziata un problema per l'Italia e non semplicemente per il Mezzogiorno. Non credo affatto - per dirla in un altro modo - che un'Italia frammentata in venti staterelli, venti Regioni che diventerebbero più o meno tutte a Statuto speciale, possa essere a quel punto un Paese realmente competitivo a livello internazionale e che questa frammentazione possa essere funzionale a chissà quale magnifica sorte dell'Italia. Da questo punto di vista, esprimo una grande preoccupazione, perché quella tesi che intende puntare su un unico motore, quello del Nord Italia, facendo sì che per sgocciolamento - si dice così

ci dicono invece che bisognerebbe puntare esattamente su una scelta diversa, e cioè avere due motori, uno al Nord e uno al Sud, e una maggiore coesione nazionale, soprattutto in una fase come quella attuale, dal *post*-pandemia che - come abbiamo ripetuto mille volte - ha accentuato gli elementi di diseguaglianza. Inoltre - lo dico davvero come una battuta, perché non ho il tempo per argomentare - c'è un altro punto che davvero ci lascia

in realtà passerebbe esclusivamente o quasi per un accordo tra il Governo centrale e le Regioni, saltando del tutto il ruolo stesso del Parlamento nazionale. Credo che questo sia completamente inaccettabile e, quindi, spero davvero che almeno su questo punto, in sede di emendamenti, si possa in qualche modo invertire questo dato e consentire al Parlamento del Paese, su un tema decisivo come quello dell'autonomia, di poter svolgere un ruolo di piena centralità e non invece il ruolo totalmente marginale al quale viene consegnato. Mi auguro che, nella maniera meno ideologica possibile, già a partire da questa mozione ma anche quando voteremo gli emendamenti, si possa avere un consenso trasversale attorno a detti temi. Colleghi, comunico che è stato depositato un ordine del giorno, a firma dei senatori Malan, Romeo, Ronzulli, Biancofiore, che è in distribuzione.

con un ordine diverso. Tutte le sperequazioni che esistono e che dico essere reali non sono conseguenza dell'autonomia differenziata che non c'è: per quel che mi riguarda, l'autonomia differenziata è lo strumento per arrivare a superare quello che invece c'è e non dovrebbe esserci in questo Paese. La mozione in discussione, dopo un'articolata esposizione in premessa da parte dei sottoscrittori, contiene otto impegni rivolti al Governo. Venendo al merito degli impegni, vorrei provare a rispondere punto per punto. In ragione del contenuto della mozione dovrò formulare anche valutazioni sull'Atto Senato 615, sebbene al di fuori del procedimento legislativo nell'ambito del quale sta avvenendo l'esame. Con il primo impegno i presentatori richiedono, prima di procedere a qualsiasi trasferimento di competenze a una o più Regioni della Costituzione, ad assicurare che siano definiti ed attuati compiutamente e preventivamente tutti i livelli essenziali delle prestazioni, A questo proposito vorrei ricordare che l'Atto Senato 615 prevede già che il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, di cui all'articolo 3, può essere effettuato secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*. Ritengo, quindi, che il Governo abbia già preso una posizione sufficientemente chiara sul punto e ribadita nel *question time* della scorsa settimana. Il procedimento di definizione dei LEP è stabilito attualmente dalla legge di bilancio per il 2023

concernenti diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, che questo Ministro ha insediato a supporto dell'operazione di individuazione dei LEP e presieduto dal professor Sabino Cassese, sta chiudendo la ricognizione di tutte le funzioni amministrative statali esercitate nelle materie che sono possibili oggetto di autonomia differenziata e - secondo una scelta che questo Ministro ha condiviso - anche nelle altre non direttamente toccate dall'autonomia differenziata medesima. Per ciascuna delle funzioni interessate si sta procedendo a verificare se esse siano già toccate da LEP stabiliti dal legislatore, come ad esempio nella sanità, oppure se si ravvisi l'esigenza di fissazione di nuovi. Personalmente ritengo che l'operazione di ricostruzione che il CLEP sta facendo e che sottoporrà alla cabina di regia contribuirà a offrire un panorama affidabile di ciò che è già stato fatto e di ciò che resta da fare, così da consentire al legislatore e al Governo di compiere le scelte ritenute migliori rispetto all'obiettivo di dare corpo ai LEP e, allo stesso tempo, alle ragioni dell'autonomia; altrimenti il Paese rimane ostaggio dell'ormai noto atteggiamento del «si sarebbe potuto ben fare altrimenti». Con il secondo impegno i presentatori chiedono al Governo di favorire in sede di esame parlamentare modifiche volte a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento nella procedura di definizione delle intese, nonché della loro piena attuazione e verifica sempre e comunque preordinata al rispetto dei principi solidaristici e partecipativi previsti dalla Costituzione. Si è proposto con il disegno di legge un coinvolgimento del Parlamento nella definizione dei LEP e nella stipula delle intese fra Stato e ciascuna Regione interessata, sia in fase di negoziazione, sia in fase di approvazione. Nella parte di motivazione della mozione, i presentatori ritengono le proposte del coinvolgimento del Parlamento non adeguate. Rispetto al silenzio della Costituzione sul punto, mi sembra che le soluzioni prospettate con il disegno di legge costituiscano già un importante passo avanti. Si può ritenere che si tratti solo di un punto di partenza e che da lì sia necessario muovere per un rafforzamento ulteriore del ruolo delle Camere. Il Governo è pronto al dialogo, come sempre, su proposte costruttive. Ricordo che uno spazio importante sarà giocato dall'autonomia regolamentare delle Camere. Col terzo impegno si chiede al Governo di favorire modifiche in sede di revisione costituzionale del Titolo V, al fine di escludere che alcune materie possano essere oggetto di autonomia differenziata. Appare singolare invero che si chieda al Governo, nel momento in cui dà piena attuazione a una disposizione costituzionale che attende dal 2001 di essere resa operativa, di modificare quelle stesse norme che lo stesso Governo e il Parlamento dovrebbero attuare. Escludere alcune materie in principio e in astratto non è una scelta condivisibile. È nella considerazione di ciascuna materia che Governo, Parlamento e Regioni interessate nel negoziato decideranno se ed entro quali limiti alcune materie saranno oggetto dell'intesa. Evidentemente, non tutte le materie interessate potranno essere devolute così, *sic e simpliciter*: saranno il negoziato, la prassi e la razionalità a definire i limiti da osservare. Con il quarto impegno si chiede di adottare misure concrete per il riequilibrio tra le Regioni e il superamento dei divari, attraverso un piano di sviluppo per le aree economicamente più svantaggiate. Si tratta di un argomento che, com'è ovvio, è condivisibile, ma che parte da un assunto che, al contrario, condivisibile non è. Tale assunto è che l'autonomia differenziata di cui all'articolo 116 sia in realtà un fattore destinato ad aggravare o a cristallizzare gli squilibri già oggi presenti nel Paese. È convinzione del Governo che l'autonomia differenziata sia esattamente una risposta efficace che i territori regionali cercano per conseguire proprio quell'obiettivo di riequilibrio, sfruttando le leve di sviluppo presenti in ciascuna comunità. Su questa premessa, voglio però rassicurare che il ruolo dello Stato non viene meno, sia nella garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), sia negli interventi perequativi ordinari e straordinari. Se si presta attenzione, è proprio nel momento in cui si discute di ampliare l'autonomia dei territori che il ruolo dello Stato è stato maggiormente interpellato. Lo stiamo vedendo proprio in questi giorni: prima dell'autonomia differenziata, il ruolo dello Stato nella definizione dei LEP era così invocato? Onestamente, bisogna rispondere di no e questo lo ritengo già un effetto positivo dell'autonomia. Con il quinto impegno, si chiede di favorire modifiche in sede parlamentare atte a garantire che l'articolo 10, comma 2, del disegno di legge non sia in contrasto con il dettato costituzionale. Si ritiene che il richiamo all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 possa costituire un buon punto di mediazione fra le diverse esigenze con l'intenzione specifica di dare alle Regioni a Statuto speciale quei margini aggiuntivi di autonomia che vengono riconosciuti alle altre Regioni. Con il sesto impegno, i presentatori chiedono al Governo di subordinare l'adozione di schemi dei con cui saranno determinati i LEP alla preventiva istituzione nella prossima legge di bilancio per il triennio 2024-2026 di un fondo di perequazione per i territori con minor capacità fiscale per abitante, da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai LEP fissati in piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali. Si tratta di un'esigenza da più parti sollecitata e che il Governo e questo Ministro condividono profondamente, se non altro per esser stato fra i proponenti, all'epoca, della legge n. 42 del 2009. Indubbiamente, l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, richiederà un'accelerazione verso la completa attuazione dell'articolo 119, anche a proposito dei fondi perequativi che sono già previsti dalla legge, ma non ancora pienamente funzionanti, a partire da quello previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Il tema della perequazione ordinaria potrà trovare compiuta assunzione nell'ambito del disegno di legge di delega fiscale ora all'esame del Senato. Con il settimo impegno si chiede al Governo di prevedere verifiche obbligatorie e costanti sull'attuazione delle intese, secondo parametri precisi, stabiliti dalla legge e con pieno coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche in possesso delle opportune competenze, eccetera. Anche a questo proposito mi sarà consentito sottolineare come spetterà a ciascuna intesa e alle leggi approvative di ciascuna intesa indicare le forme di monitoraggio più efficaci sull'attuazione delle intese medesime, sulla base di quanto previsto dalla legge generale di attuazione. Vorrei ricordare infatti che il tema è già affrontato dall'articolo 7 dell'Atto Senato 615. Rilevanti affinamenti e precisazioni sul tema del monitoraggio sono contenuti in emendamenti appena presentati da Gruppi di maggioranza, in consonanza con non pochi emendamenti dei Gruppi di opposizione. Da ultimo, c'è l'ottavo impegno, con cui si chiede al Governo di monitorare gli effetti della differenziazione su tutte le Regioni. Da una parte l'impegno al monitoraggio non solo è condivisibile, ma è pure doveroso, proprio nell'esercizio del ruolo dello Stato. La finalità del disegno di legge n. 615 è proprio quella di contrastare la frammentazione e la duplicazione delle funzioni. Anche a questo riguardo sono state condivise alcune proposte migliorative, al fine di assicurare la verifica dell'effettività dei LEP anche nelle Regioni estranee alle intese, prevedere verifiche sui profili finanziari da parte di organismi terzi, disciplinare le ipotesi di modifica o cessazione anticipata delle intese, confermare l'applicazione dei poteri sostitutivi statali, di cui all'articolo 120. Concludendo, ringrazio i presentatori per l'affezione dimostrata nei confronti del disegno di legge n. 615, che è spesso oggetto di *question time*, sia alla Camera dei deputati Sono molto soddisfatto delle 60 audizioni che abbiamo svolto in Commissione, dei quasi 50 interventi in discussione generale, delle due settimane di presentazione e illustrazione degli oltre 570 emendamenti. Fare di più è sempre meglio e possibile, però qualche volta il meglio è nemico del bene. Sollecito tutti, oltre alla discussione delle mozioni,

Sugli impegni, esprimo parere contrario al primo impegno, parere favorevole sul secondo impegno e parere contrario al terzo impegno. parere favorevole con la seguente riformulazione: «ad adottare misure concrete per il riequilibrio tra le Regioni e il superamento dei divari esistenti, in attuazione dell'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma della Costituzione».

«a favorire, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge Atto Senato 615, modifiche volte a rafforzare i meccanismi di verifica sull'attuazione delle intese, assicurando il pieno coinvolgimento delle istituzioni pubbliche in possesso delle opportune competenze, al fine di garantire, sull'intero territorio nazionale, l'effettività dei principi di solidarietà territoriale e coesione sociale». Sull'ottavo impegno, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «a favorire, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge Atto Senato 615, modifiche volte a prevedere forme di monitoraggio degli effetti della differenziazione su tutte le Regioni, non solo quelle con le quali si raggiunge l'intesa, anche al fine di prevenire fenomeni di frammentazione amministrativa e normativa e duplicazione degli enti». Il testo delle riformulazioni è stato

Peraltro, avrà visto che questa è una mozione firmata non solo dal mio Gruppo, ma anche da senatori di altri Gruppi quindi è bene che ci sia un minimo di approfondimento.

risponda a verità il fatto che, in sede di Conferenza dei Capigruppo, si fosse convenuto di limitarsi esclusivamente alle dichiarazioni di voto e non procedere alla presentazione di singoli ordini del giorno.

Signor Presidente, nella Conferenza dei Capigruppo non abbiamo convenuto sul fatto di poter abbinare delle mozioni come si fa generalmente, secondo la prassi. Questo non è stato convenuto. La possibilità di presentare ordini del giorno è prevista dal nostro Regolamento. [DE

cioè la modifica costituzionale volta a realizzare la massima forma di democrazia attraverso l'espressione diretta della volontà popolare: il presidenzialismo o premierato nelle declinazioni di cui si sta discutendo.

c'è un partito di maggioranza, Fratelli d'Italia, che non lo può dire ma è evidentemente in grande difficoltà su un tema come quello dell'autonomia differenziata,

Il combinato disposto di queste due posizioni è esattamente l'accordo politico al quale stiamo assistendo: io ti do l'autonomia differenziata e in cambio ti do il premierato. Tu prendi il premierato e in cambio ti silenzi sull'autonomia differenziata.

adesso; queste due rilevantissime questioni - il presidenzialismo o il premierato, da una parte, e l'autonomia differenziata, dall'altra - non sono due argomenti serissimi che si stanno discutendo nel merito, uno separatamente dall'altro, affrontandone gli elementi positivi e quelli negativi,

oggettivamente bisogno di un approfondimento per essere comprese, ma anche, come è stato anticipato, per la presentazione, diciamo così, a sorpresa di questo ordine del giorno che mette nero su bianco i sospetti che aleggiavano intorno a questo progetto fin dall'inizio. Adesso i sospetti sono diventati assolutamente realtà e sono leggibili a tutti, all'Assemblea e anche al Paese. Siamo di fronte ad un autentico scambio politico. L'autonomia differenziata per la Lega, indigesta per Fratelli d'Italia,

È davvero sconcertante che si sia deciso di scoprire le carte così, mostrando anche una debolezza interna alle forze di maggioranza. Il mio Gruppo chiede allora un momento di approfondimento anche per capire, visto che ci sono state versioni contrastanti,

si stia trasformando in un'altra occasione perduta. Lo dico per i colleghi e le colleghe che nella Conferenza dei Capigruppo sono rappresentati da tutti noi presidenti dei Gruppi. In quella Conferenza, Presidente, noi abbiamo deciso di non seguire il Regolamento per consentire a questa giornata di essere caratterizzata da un confronto sulle nove mozioni; per questa ragione non c'è stata, presidente Romeo, discussione generale e, sempre per questa ragione, non poteva essere presentato, come dice il Regolamento, un ordine del giorno al termine della discussione generale, perché essa non c'è Tutti noi, rappresentanti dei Gruppi di opposizione, avevamo rigorosamente deciso di non presentare ordini del giorno e lo avevamo fatto rispettando una sorta di *gentlemen agreement* che era stato raggiunto perché volevamo discutere del merito delle mozioni. Tra l'altro, ministro Calderoli, non è un caso che mozioni su nove, probabilmente potrebbero uscire da quest'Aula con una larghissima maggioranza e nessuno ha guardato i programmi

venga qui in Aula, smonti una sola mozione, pezzo per pezzo, provando a rifare un passaggio che era già avvenuto in Commissione affari costituzionali, dicendo di fatto all'Assemblea può dire quello che vuole, tanto alla fine decide lui perché questo è il programma di Governo - lo dico ai colleghi della maggioranza - rischia di far saltare la giornata che avevamo costruito. signora Presidente, chiedo la sospensione dei lavori perché non erano queste le regole del gioco e chiedo ai colleghi della maggioranza di non presentare - e se l'hanno già fatto di ritirarlo - quell'ordine del giorno. Democraticamente l'Assemblea si esprimerà sulla mozione a prima firma del senatore De Cristofaro, che probabilmente sarà respinta, come è normale che sia nel gioco democratico, ma quello che non possiamo consentire - lo dico non tanto per oggi, quanto per la prosecuzione dei nostri lavori e dei nostri rapporti

voglio chiarire una cosa: sia l'autonomia differenziata, sia una riforma volta a dare maggiore peso all'indicazione degli elettori rispetto al Capo dell'Esecutivo sono contenute nel programma comune a tutte le forze del centrodestra.

Poiché mi sembra che più che contestare il metodo, essendo conservata la facoltà di depositare un ordine del giorno, si contesti anche il merito di questo ordine del giorno, mi riservo di sentire la Presidenza e quindi sospendo la seduta per venti minuti.

16 luglio 2023, presso il *terminal* A dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania, si è sviluppato un incendio che da quello che è emerso e da informazioni frammentarie (certezze non ne abbiamo da nessuno, perché la vicenda si connota per una fumosità anche delle informazioni oltre che dell'incendio in sé), sarebbe stato causato dal malfunzionamento di uno degli impianti di condizionamento dell'aria. La società che gestisce l'aeroporto ha gestito questa emergenza con un

cui sembrava che avrebbe ripreso ad operare il 25 luglio. È notizia delle ultime ore che probabilmente se ne parlerà non prima dell'inizio di agosto; inoltre, anche in questo caso non abbiamo nessuna certezza, quindi continuiamo a rimanere in questo stato di approssimazione e di assoluta incertezza su quello che accade all'aeroporto. Presidente, l'aeroporto di Catania, Vincenzo Bellini, è il primo scalo internazionale della Regione Siciliana, ma è anche uno dei più grandi aeroporti e scali internazionali d'Italia. allora che un aeroporto chiuda per un qualsiasi motivo - tra l'altro osservo che il Vincenzo Bellini non è nuovo a chiusure, anche temporanee, per i fenomeni eruttivi dell'Etna, che spesso, con le ceneri che si disperdono nell'aria, causano la necessità di interrompere i voli

Questa considerazione, però, non è fine a se stessa e men che mai può essere considerata come una mera lamentela di una cittadina siciliana. Al contrario, è veramente

del Presidente)*. Quello che infatti è emerso dalla gestione di questa emergenza è, innanzitutto, un danno incalcolabile per la Regione Sicilia, per il suo turismo, per la sua economia, per lo stato dei servizi degli stessi cittadini siciliani. Non sappiamo quando riprenderanno i voli;

dell'incendio della discarica di Bellolampo, i cui fumi hanno reso impraticabile l'aeroporto per tutta la mattinata. Allora, se i due scali fondamentali dell'isola chiudono o hanno necessità di chiudere per qualche ora, com'è successo anche a Palermo, è inimmaginabile che non ci sia un piano di gestione delle emergenze, cioè che non si sappia, in caso di chiusura di uno dei due scali

colleghi, chi deve partire da Catania per raggiungere una destinazione non sa se riuscirà a partire da Catania o se, raggiunto l'aeroporto di Catania, non verrà messo su un pullman per raggiungere Comiso o Trapani e partire da lì; viceversa, chi aveva già prenotato voli con atterraggio su Catania non sa se atterrerà su Catania o se, invece, atterrerà su Comiso

era pensato di godere in Sicilia e che sono saltate, per quelle famiglie che avevano messo da parte i risparmi per trascorrere un'esperienza in Sicilia. È un danno incalcolabile anche per l'immagine della Sicilia, che appare sempre di più come una terra, non soltanto desolata

sia necessario avviare un'indagine - lo chiedo con forza al Governo -perché si deve sapere che cosa è successo, ma soprattutto si devono capire quali sono state le criticità e le inefficienze di un sistema che evidentemente non ha saputo gestire un'emergenza. Chiedo altresì che venga adottato

un territorio collegato stabilmente con il resto dell'Italia e dell'Europa. Occorre dunque potenziare i mezzi di trasporto per raggiungere l'aeroporto di Reggio Calabria, soprattutto se, come ha dichiarato il Ministro dei trasporti, le limitazioni sull'aeroporto verranno eliminate per cui diventerà finalmente uno scalo attrattivo e capace di gestire l'area conurbata di Messina e di Reggio Calabria.

Signor Presidente, innanzi tutto voglio ringraziare la collega Musolino, perché ha sollevato una questione che oggettivamente sta creando notevoli difficoltà a quel territorio; lo ha fatto con competenza e individuando soluzioni che - me lo faccia dire, signor Presidente - probabilmente, molto probabilmente, avrebbero già dovuto essere oggetto di un'iniziativa da parte del ministro Salvini.

e gli aeroporti, per diverse ragioni, stanno collassando. Non c'è mai stata nella storia di questo Paese una situazione di tale gravità e difficoltà nel bel mezzo di un momento turisticamente delicato per tutti noi. Ribadisco che viviamo una stagione di rinascita dal punto di vista turistico dopo l'emergenza Covid, che tutti avevamo auspicato fosse davvero di ripresa e alla quale avevamo tutti immaginato di arrivare pronti e con le capacità che il nostro sistema è in grado di mettere in campo. E invece,

abbiamo una situazione complessiva che fa davvero venire i brividi in termini di biglietto da visita che stiamo dando al resto del mondo sulla vocazione principale del nostro Paese. E cosa fa il ministro Salvini? Va a parlare di tutt'altro e intanto ci sta ancora raccontando che realizzerà in tempi rapidissimi il ponte sullo Stretto di Messina. Noi ovviamente siamo a favore

maturare una qualche perplessità rispetto alla capacità di realizzazione di una delle opere più difficili e imponenti che ci saranno al mondo. Naturalmente, abbiamo sempre detto di essere a disposizione essere a disposizione di chi vuole fare, però siamo anche quelli che denunciano quando le cose non si fanno. Faccio un esempio molto chiaro: in queste ore, sul versante del territorio ligure, ma anche lombardo, abbiamo una situazione di grave difficoltà della rete infrastrutturale, anche dal punto di vista stradale. La Gronda è bloccata (si dice che non ci siano i soldi); la TAV non mi pare che abbia fatto grandi passi in avanti (non so se la collega Fregolent ha visto qualche metro in più di realizzazione dell'opera, ma non mi risulta, visto che è molto attenta a quell'intervento, così come il collega Borghi). Abbiamo quindi una situazione di stallo complessivo delle infrastrutture. A fronte di ciò, non riuscite a utilizzare

rimane diviso a metà a ogni pioggia e a ogni grandinata. Questa è la verità sul Governo della realizzazione, sul Governo di chi doveva essere pronto e sul rimpallo di responsabilità indecente che abbiamo visto nei giorni scorsi tra il ministro Urso e il ministro Salvini. Un rimpallo di responsabilità che oggi ha portato la collega Musolino a chiedere che, in realtà, il problema venga risolto a livello regionale. Abbiamo due Ministri, abbiamo un Presidente di Regione il dato di fatto è che quell'aeroporto è ancora chiuso, compromettendo moltissimo il turismo in una Regione fondamentale per il PIL del Paese. la motivazione con la quale voteremo molto volentieri la mozione portata avanti dalla collega Musolino. Ci fa piacere che anche il Governo, in qualche modo, abbia dato l'*ok*. Evidentemente le nostre denunce sono vere e state continuando a fare una graditissima autocritica. la mozione Musolino affronta oggi un tema di forte attualità, che riguarda la nostra Sicilia. Si tratta davvero di una situazione surreale, che sta generando un danno all'immagine e soprattutto alla qualità del servizio della nostra terra. servizio aereo è veramente allo sbando in questo momento, anche perché stamattina è stato chiuso l'aeroporto di Punta Raisi, a causa di un incendio nelle zone limitrofe. Quindi la situazione è davvero grave. L'aeroporto di Catania sta diventando di giorno in giorno sempre più insostenibile, signor Sottosegretario, una vera e propria bomba bomba ad orologeria, che si riflette anche sugli altri scali siciliani, perché non si è ben organizzati e non si è ben strutturati per poter accogliere, oppure per poter effettuare le partenze. Esprimo però orgoglio, poiché la mozione della senatrice Musolino è stata accolta con parere favorevole da parte del Governo. Certamente la SAC, la società che ha in gestione l'aeroporto di Catania, deve dare delle risposte su una più puntuale programmazione della manutenzione, sulle verifiche infrastrutturali e delle infrastrutture stesse. Ora risultano essere al lavoro cinque aziende, impegnate con più squadre nei lavori di pulizia e bonifica al *terminal* A dell'aeroporto di Catania, per farlo tornare in piena attività operativa. Tra loro c'è anche una società specializzata nel ripristino dopo incendi, che ha già lavorato sul *terminal* 3 di Fiumicino, dopo l'incendio del 2015. Certamente bisogna ripristinare la situazione di operatività degli scali siciliani, come ho detto poc'anzi, in un periodo di altissima stagione, con le strutture ricettive che sono piene di turisti. turisti. Bisogna evitare danni al sistema produttivo di Catania e della Sicilia orientale, causati dal blocco dei voli e dalla perdita di reputazione dell'aeroporto stesso. Quindi ci auguriamo che venga ripristinata al più presto la piena operatività dell'aeroporto. Va ricordato che la Sicilia è un'isola e, senza i suoi aeroporti, muoversi diventa davvero molto difficile. Peraltro bisogna garantire ai cittadini la continuità territoriale per collegare l'isola al continente e l'incidente ha reso quanto mai attuale la necessità di avviare un piano di investimenti per adeguare le infrastrutture alle esigenze del territorio a livelli europei.

Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, quello che è accaduto il 17 luglio è, come si suol dire, l'ulteriore riprova che il Governo dei migliori, quelli bravi, quelli pronti, non era ancora una volta pronto a risolvere i problemi reali che i cittadini vivono. verificato un incidente in una piccola porzione dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, uno scalo di interesse internazionale con un potenziale enorme, che però negli ultimi anni, almeno una decina, non riesce a mettere a terra tutti quelli che sono i progetti e i piani di ampliamento e adeguamento. La questione non è limitata o localizzata al problema dell'aerostazione Fontanarossa di Catania. Ciò ha fatto emergere in maniera palese, chiara ed inequivocabile che all'interno della Regione Siciliana c'è chi non riesce a programmare in maniera adeguata adeguata il miglioramento di quello che è tutto il sistema intermodale e dei trasporti dell'isola. Qual è il paradosso dei paradossi? Vado

che ha vinto anche il bando di gestione dell'aeroporto di Comiso, continui - non so secondo quali logiche, dinamiche o fini oscuri, almeno a me - a tenere sotto scacco tutta quell'area, senza potenziare l'aerostazione o riuscire ad organizzare una gestione adeguata ed ottimale, anche utilizzando lo scalo dell'aeroporto Magliocco, di

rimedio fino a quando la società stessa possa mettere a terra il progetto del grande aeroporto internazionale di Catania. Abbiamo già proposto anche al Ministro, all'uomo del Ponte, di provvedere nel giro di poco tempo, almeno a potenziare la rete raddoppiando gli Intercity per Roma e per Milano, sgravando al contempo il grande traffico legato anche agli scali di Napoli, Roma, Pisa e Milano.

il tema del trasporto aereo e dal collegamento delle isole sarà importantissimo. Abbiamo inserito nella scorsa legislatura anche il tema dell'insularità in Costituzione e dobbiamo essere consequenziali.

Signor Presidente, nell'ascoltare gli interventi dei rappresentanti delle opposizioni, mi sono incuriosito di questa nuova modalità modalità molto generalista di affrontare i problemi del Paese; un po' quello che è accaduto prima mentre il ministro Calderoli stava tentando di spiegare principi e criteri di funzionamento del nuovo progetto di responsabilizzazione dei territori. Qui siamo in una situazione più o meno paritetica e mi dispiace che quello che qualcuno prima chiamava l'uomo del Ponte, cioè il ministro Matteo Salvini, pochi giorni fa abbia spiegato tecnicamente che cosa significa gestire un aeroporto e quali siano le responsabilità alle quali è chiaramente chiamato il soggetto tenuto a gestire una struttura aeroportuale. Il gestore aeroportuale, con tecnica e perizia, dovrebbe garantire l'efficienza e l'operatività dell'aeroporto stesso,

ci sia una prevenzione rispetto agli incidenti, ma anche per superare le situazioni di crisi. In particolare, l'aeroporti di Catania è affidato - lo si ricordava prima - ad una società per azioni partecipata da vari soggetti pubblici. Nello specifico, ci troviamo chiaramente d'accordo con i contenuti e con le conclusioni della mozione che è stata presentata. Certamente un'indagine ispettiva - guarda caso - è quello che in altra maniera il ministro Salvini poche ore fa ha

con le dovute differenze, sono gestiti come le spiagge: c'è un bando di gara e c'è un soggetto che ha la responsabilità di gestire, attraverso un titolo concessorio. In particolare dopo il rogo del 16 luglio, come sappiamo, nel *terminal* A si sono verificate delle cancellazioni e si sono purtroppo dovuti dirottare dei voli su altri scali e in questa occasione si è parlato del potenziamento, ad esempio, dell'altro aeroporto importante nella limitrofa Regione Non posso ovviamente non ricordare le parole che sono state usate poco fa e lo vorrei fare cercando invece di chiarire quello che il MIT ha espresso chiaramente, con l'obiettivo di accelerare il ritorno alla normalità. Da parte del Ministro è stato confermato il pieno spirito collaborativo, anche se

di questo tipo di eventi. Vorrei anche ricordare - forse nessuno l'ha ancora detto - che quello di Catania è un aeroporto particolare anche per una situazione un po' unica al mondo, ovvero quella di trovarsi accanto a un vulcano che spesso determina

peraltro riconosciamo assolutamente l'esigenza di rivedere il sistema aeroportuale del Sud potenziandolo. In questo siamo vicini al ministro Salvini, che ha anticipato la sua disponibilità per venire incontro alle difficoltà mostrate dalla società che ha in gestione l'aeroporto. siamo molto contenti della disponibilità del ministro Salvini a occuparsi del tema, ma va detto che in alcuni casi ci sono dei doveri e non soltanto delle disponibilità. Piacevolmente, peraltro, abbiamo anticipato in diverse interrogazioni la necessità di occuparsi sia delle questioni di emergenza dell'aeroporto di Catania, sia precedentemente della questione del caro voli che riguarda soprattutto la Sicilia. La Sicilia è un'isola. Questo significa avere la consapevolezza di quanto costano le alternative, di come si vive, di come si soddisfano i bisogni essenziali quando basta un piccolo evento a generare un'enorme fragilità. Noi veniamo da ventiquattr'ore nelle quali a Palermo una donna è morta perché non ha potuto essere soccorsa a seguito degli incendi; l'aeroporto di Palermo è stato chiuso per alcune ore; stamattina l'aeroporto di Catania era Catania era attrezzato, peraltro con una ottima disponibilità del personale che va a ringraziato, come se fosse un momento di grandi vaccinazioni, un momento pandemico, un momento di emergenza, di grande caos. Tutto questo esattamente nel momento in cui il turismo è al pieno della sua forza, della sua onda, e nel momento in cui tante persone partono dalla Sicilia e vengono in Sicilia magari con alcuni risparmi, dato il fatto che questi voli costano così tanto, per fare qualche giorno di vacanza. Cito tre storie che mi sono arrivate: la prima è quella di Omar, che ha il problema che ormai il ritardo che è stato generato nel suo itinerario di viaggio gli rende molto più costoso il viaggio per cui vorrebbe rinunciarvi; tuttavia nello stesso tempo gli hanno detto che se cancella il volo gli potrebbero essere attribuite delle penali; alla fine, quindi, sta decidendo di partire nonostante abbia dei costi per ridurre gli extracosti che la rinuncia al viaggio gli comporterebbe. Un gruppo di turisti inglesi si è trovato ad atterrare a Trapani anziché a Catania; sono usciti per cercare una navetta, hanno visto delle navette che stavano a mare, ma nessuno li ha informati che si trovavano in un'altra città. A Palermo è successa la stessa cosa: alcuni personaggi hanno offerto viaggi privati da Palermo a Catania con dei costi molto esosi. Questo significa oggi essere in Sicilia quando

La Sicilia è il luogo nel quale la Presidente del Consiglio, il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno avuto l'offerta di dirette televisive in occasione delle scorse elezioni amministrative, ma quando c'è da affrontare con urgenza questi temi occorre farlo. C'è bisogno di istituire un fondo adesso, c'è bisogno di dare soccorso alle persone che hanno avuto danni alle infrastrutture, alle imprese, agli stessi cittadini che hanno bisogno di essere rimborsati, ma ciò non sta avvenendo. Noi siamo d'accordo con l'idea che debba esserci un piano di emergenza che sia operativo per tutte le emergenze che riguardano la mobilità in Sicilia e non soltanto gli aeroporti, tuttavia vorremmo anche chiederci se dobbiamo applicare alla questione siciliana il parametro che questa mattina la

ad approvare questo piano. Mi verrebbe in mente il titolo di un romanzo di un siciliano, Leonardo Sciascia, intitolato «A ciascuno il suo», ma preferisco un altro suo romanzo da un titolo evocativo, «La Sicilia come metafora». Non vorremmo che il disastro che la Destra sta realizzando in Sicilia si estenda man mano al resto del Paese. Non ne abbiamo bisogno; abbiamo invece bisogno di interventi seri, di impegni concreti. La Sicilia in particolare è in grandissima difficoltà in queste ore. Serve uno sforzo, un impegno finanziario importante di questo Governo, un sostegno significativo perché si stanno realizzando danni complessivi che interessano i cittadini siciliani, ma anche i cittadini che hanno scelto

Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, la mozione presentata dalla collega Musolino credo abbia l'indiscusso merito di affrontare una tematica di grande attualità e molto delicata, quale certamente è quella dell'incendio che si è verificato il 16 luglio scorso presso il *terminal* arrivi dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. Un evento assolutamente imprevisto e imprevedibile, che ha determinato enormi disagi a centinaia di migliaia di passeggeri, con il contestuale enorme danno economico arrecato al sistema economico-produttivo della nostra Regione, in particolare al comparto turistico, che in questi ultimi anni ha registrato un tasso di crescita a doppia cifra, con un *record* assoluto di arrivi e di pernottamenti. Vincenzo Bellini - come è stato ricordato - è il quinto aeroporto italiano, con oltre 10 milioni di passeggeri, e in questo periodo vedeva transitare oltre 40.000 passeggeri al giorno. Non sta a me certamente attribuire eventuali responsabilità, anche perché è in corso un'inchiesta della procura etnea; ma con la stessa franchezza dobbiamo dire che qualcosa evidentemente non ha funzionato anche se non è questo né il momento, né il luogo all'interno del quale potersi confrontare su questa tematica. Questa vicenda ha altresì evidenziato - lo dobbiamo dire con chiarezza - la fragilità del sistema infrastrutturale siciliano, all'interno di un contesto in cui con altrettanta schiettezza dobbiamo dire che si registrano nette inversioni di rotta, laddove il Governo Meloni, il ministro Salvini e il vice ministro Bignami hanno puntualmente esternato un progetto di miglioramento infrastrutturale della nostra Regione, che riguarda 28 miliardi di euro (contrariamente a quello che ha detto il mio amico e collega Nicita). Penso agli investimenti sulla rete ferroviaria Messina-Catania-Palermo di 10,8 miliardi; penso alla metropolitana di Catania, che arriverà all'aeroporto e che arriverà altresì altresì fino a Paternò e a Adrano; penso alla Catania-Ragusa da 1,5 miliardi di euro; penso altresì al Ponte sullo Stretto, che finirà di rappresentare il sogno proibito dei siciliani. Quanto accaduto credo abbia evidenziato l'assoluta necessità di nuovi investimenti infrastrutturali all'interno dell'aeroporto di Catania, ma credo di poter dire, senza timore di smentita, che abbia evidenziato anche l'assoluta necessità di investimenti aggiuntivi all'interno dell'aeroporto di Comiso, che - come il collega Sallemi sa meglio di altri può svolgere una funzione fondamentale all'interno del sistema infrastrutturale della Sicilia sudorientale, anche alla luce di alcune peculiarità presenti all'interno dello scalo etneo, laddove i fenomeni eruttivi dell'Etna talvolta ne determinano la chiusura. Mi auguro quindi che si possa tornare gradualmente alla normalità, grazie anche alla sinergia tra Governo nazionale e con il governo regionale. Preannunzio pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

Colleghi, riprendiamo l'esame della mozione relativa alla candidatura di Roma come città ospite di Expo 2030, sulla quale c'erano già stati tutti gli interventi e che dobbiamo solo mettere in votazione. votazione. Vi ricordo che c'è un parere favorevole del Governo, con espunzione del terzo impegno, così come proposto dal presentatore De Priamo.

costante che, come Italia Viva e Azione, abbiamo sempre fatto in questi mesi in maniera propositiva sulla sanità. Una sanità pubblica italiana che, nonostante tutte le difficoltà, è ancora oggi un fiore all'occhiello in Europa e nel mondo, un modello di tutela universale della salute. *(Brusio).* Signor Presidente, potrei chiedere per favore un po' di silenzio? È

Dicevo che la sanità pubblica, come sappiamo, sta incontrando notevoli difficoltà, soprattutto dopo il Covid e per il divario sempre più crescente tra Regioni e tra aree geografiche, ma soprattutto perché è andata in difficoltà - a causa della carenza di medici, di infermieri, di tutto il personale sanitario - la medicina territoriale, la medicina di base.

basta guardare i dati, andare in qualsiasi ospedale o pronto soccorso per capire quello che sta accadendo, leggere l'osservatorio o il rapporto di cittadinanza attiva, dove si dice che addirittura il 40 per cento degli italiani ha rinunciato allo *screening*: è una cosa gravissima e vuol dire che salta tutto il sistema della prevenzione. Mi vorrei concentrare anche sulle proposte, perché purtroppo - ahimè - conosciamo quali sono i dati drammatici che ho appena elencato. Le proposte sono quelle di reperire risorse finanziarie necessarie a rispondere alla criticità che ho richiamato in premessa; ad adottare iniziative volte a favorire il ricambio generazionale del personale medico e infermieristico; ad intervenire per assicurare per assicurare maggiori attrattività alle professioni sanitarie incrementando le remunerazioni e le indennità specifiche; ad elaborare finalmente un piano nazionale pluriennale di interventi di prevenzione; a prevedere anche un piano un piano di potenziamento della sanità e assistenza territoriale; ad adottare anche un piano nazionale di edilizia ospedaliera, sapendo

che vuole contrastare il dilagare continuo di *fake news* e di posizioni antiscientifiche, che abbiamo già visto durante la pandemia e che però, purtroppo, continuano a destabilizzare e a creare un clima di sfiducia anche nei confronti delle istituzioni. ad adottare iniziative volte a contrastare la continua fuga di cervelli anche in ambito sanitario e, al contempo, incentivare forme di valorizzazione e attrazione di talenti anche dall'estero; Negli ultimi otto anni il 41 per cento dei nostri migliori cervelli (scienziati, ricercatori, medici) è andato all'estero, ma non per studi: sono andati all'estero con un alto livello di istruzione e poi sono rimasti lì, dove hanno hanno avuto sicuramente maggiori remunerazioni, soddisfazioni e riconoscimenti nell'ambito del proprio lavoro. Anche su questo chiediamo al Governo, dunque, un impegno ben preciso per valorizzare questi cervelli, attraendo però anche tanti talenti che provengono dall'estero, perché sappiamo che, all'interno dell'Unione europea, siamo il Paese che attrae meno scienziati e ricercatori provenienti da altri Stati. a garantire la piena ed efficace implementazione del fondo di cui all'articolo 104, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 34, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, per consentire l'erogazione degli ausili e delle protesi degli arti inferiori e superiori: si chiede quindi di consentire di inserire anche questa parte, aggiornando i LEA e tutte le prestazioni che necessitano ovviamente di un aggiornamento sistematico e periodico del nomenclatore.

un amore per il Servizio sanitario nazionale pubblico, che ritengo essere un valore uniformemente condiviso sicuramente dalla maggioranza, ma anche dell'opposizione. Su questi temi non ci si deve dividere, ci si deve unire. Verrebbe facile ora, richiamando le parole della collega, alla quale mi lega anche un affetto frequentando la stessa Commissione, parlare di una filiera di responsabilità, che evidentemente non pongo in campo. Noi governiamo da sei mesi e il Sistema sanitario nazionale pubblico

cito sempre, come prima esperienza da parlamentare, l'anno 2018, anno in cui il fondo sanitario nazionale si dotava di 114 miliardi di euro. La fondazione GIMBE, mai parca di complimenti nei confronti della maggioranza del centrodestra - ben vengano le critiche costruttive - racconta che nel 2018, nei dieci anni precedenti, erano stati definanziati 37 miliardi di euro al fondo sanitario nazionale; un dato importante dal quale partire anche per argomentare e quindi per trovare insieme le soluzioni. C'è stato poi il Covid ed è stato implementato il fondo sanitario nazionale proprio per rispondere a tutta una serie di esigenze legate all'acquisto delle mascherine e dei vaccini e all'assunzione di personale sanitario. Bene:

Cito questi dati *per tabulas*, proprio per aprire anche al dibattito conseguente a queste mozioni, perché ritengo che la centralità del Senato e di tutte e due le Camere del nostro Parlamento sia fondamentale, come lo è riportare verità e numeri. I numeri nel loro essere asettici

Ma è evidente che, se lo parametriamo all'economia durante il Covid, essendo il coefficiente un rapporto fra un numeratore e un denominatore

ricordare - il Governo Meloni non ha fatto altro che ripercorrere dati e cifre che erano stati presentati l'anno precedente dal precedente Governo. quindi si grida allo scandalo rispetto a un presunto definanziamento del fondo sanitario nazionale rispetto al PIL, vi invito a leggere la relazione al DEF del precedente Governo, che è sovrapponibile a quella del Governo Meloni, con una differenza, però: mentre si redigeva quel documento, c'era tecnicamente ancora il Covid; quando invece il Governo Meloni ha posto mano al DEF, e quindi finanziato per i tre anni successivi il fondo sanitario nazionale, per nome e quindi per intervento del presidente dell'OMS, il dottor Tedros Ghebreyesus, si sancisce che il Covid non c'è più.

tutto quanto previsto rispetto alla programmazione sanitaria: vi registro infatti che, se oggi non abbiamo medici o infermieri, banalmente è il risultato di una cattiva programmazione fatta dieci anni fa; un medico può esercitare in Italia - tranne le ultime le ultime modifiche apportate durante il Covid e da noi comunque confermate - solo se è laureato in medicina e, quindi, ha fatto un percorso di studi di sei anni e ha conseguito una specializzazione (mediamente, altri quattro anni). Se oggi decidiamo - così come abbiamo fatto

anni. Se oggi ci troviamo quindi in penuria di medici, lo registriamo, ma per amor di verità diciamo che sostanzialmente tutto questo è avvenuto quando evidentemente la programmazione era stata fatta Mi premeva dire questo e ora lo faccio in maniera veramente sommessa, ma premettendo che la validazione dell'articolo 32 della nostra Costituzione non dev'essere patrimonio del centrodestra o del centrosinistra. Deve essere patrimonio comune del Parlamento e comune a chiunque venga eletto

Rispetto alle premesse, il Governo esprime parere contrario. Per quanto riguarda gli impegni, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: «valutare ogni altra iniziativa utile a reperire le risorse finanziarie necessarie a rispondere alle criticità richiamate, volte in particolare a sostenere il finanziamento del sistema sanitario sul breve, medio e lungo periodo, favorendo gli incrementi dell'organico medico e infermieristico e contribuendo alla riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche e per interventi terapeutici e assistenziali riabilitativi e a non pregiudicare direttamente il fondamentale diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione e il carattere universale del sistema sanitario nazionale nel suo complesso». Per quanto riguarda il secondo impegno, il parere è favorevole, con la seguente riformulazione: «in linea con iniziative già assunte, ad adottare iniziative volte a favorire il ricambio generazionale del personale medico e infermieristico, anche al fine di non imporre turni e ritmi di lavoro eccessivi, estenuanti e senza tregua e al contempo favorire l'aggiornamento delle professionalità operanti nel sistema sanitario nazionale, senza disperdere le esperienze acquisite e proseguendo nel già avviato percorso di stabilizzazione volto a ridurre il precariato nelle professioni sanitarie e nel sistema sanitario nazionale». impegno il parere è favorevole, con la seguente riformulazione: «a proseguire nella valutazione di interventi volti ad assicurare una maggiore attrattività delle professioni sanitarie, favorendo l'incremento delle remunerazioni e delle indennità specifiche ed il rafforzamento delle tutele contrattuali, al fine di tenere in debita considerazione le peculiarità del comparto, sia al fine di far fronte alla carenza di personale in generale, sia per evitare l'afflusso delle nuove professionalità verso specializzazioni considerate maggiormente redditizie». impegno il parere è favorevole, con la seguente riformulazione: «a proseguire ed implementare le attività delineate nel piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025, al fine di rafforzare un sistema di prevenzione già fortemente provato dalla carenza di risorse finanziarie, umane e strumentale». impegno il parere è favorevole, con la seguente riformulazione: «in coerenza con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 maggio 2022, n. 77, recante «Regolamento recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del servizio sanitario nazionale», a potenziare la sanità e l'assistenza territoriale, applicando il modello della medicina proattiva (o di iniziativa), al fine di superare la tradizionale medicina d'attesa, attraverso attraverso un'attività di pianificazione articolata e complessa, volta ad individuare e rispondere preventivamente ai bisogni ed eventuali fattori di rischio per la salute dei cittadini. impegno il parere è favorevole, con la seguente riformulazione: «proseguire ed implementare le attività rivolte al rinnovamento delle strutture sanitarie, i cui edifici risalgono, nel 70 per cento a più di cinquanta anni fa, anche al fine di rafforzare le strutture dedicate ed agevolare l'assistenza di parenti e congiunti, nonché per agevolare l'implementazione delle più avanzate tecniche mediche della medicina di precisione e personalizzata». Infine, ci sono stati tre impegni successivi, rispetto ai quali sono arrivati adesso

ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica", anche nell'ottica di un prossimo aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni che tenga conto delle finalità del predetto fondo e dei costanti progressi scientifici e della ricerca sul tema, prevedendo un aggiornamento sistematico e periodico del nomenclatore.

i dispositivi sono stati di fatto riformulati in modo molto articolato dal Governo, prima di poter esprimere un parere in modo compiuto, vorremmo avere la possibilità di leggere

Presidente, credo possiamo trovarci tutti d'accordo sul fatto che i tagli, peraltro significativi, ai finanziamenti destinati al programma di ricerca per la sanità pubblica e alla vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure non possono passare inosservati perché riguardano il nostro futuro e la nostra salute, che dovrebbe essere un diritto inviolabile. Evidenziamo inoltre, così come fa il testo della mozione a prima firma della collega Paita, l'inesistente supporto così come gli scarsi investimenti nel settore sanitario pubblico a fronte del fatto che gli stanziamenti previsti sono interamente rivolti al contrasto dell'inflazione, dei costi dell'energia, dell'acquisto dei vaccini e farmaci In questi mesi, già dall'ultima legge di bilancio, abbiamo notato una totale mancanza di prospettive per il potenziamento del sistema sanitario nonostante l'aumento della spesa pubblica durante la pandemia. Siamo d'accordo con la richiesta di reperire le opportune risorse finanziarie necessarie a rispondere alle criticità del settore sanitario evitando definanziamenti e garantendo il diritto alla salute a tutti, a cominciare dal rinnovo contrattuale per tutto il personale sanitario, mettendo fine a quella spirale di precarietà che purtroppo caratterizza non soltanto la sanità, ma anche ad esempio l'istruzione. È necessario mettere a punto un piano nazionale di prevenzione e di assistenza territoriale, con un'attenzione alla medicina proattiva e avviare un piano nazionale di edilizia ospedaliera per rinnovare le strutture sanitarie e agevolare l'implementazione di tecniche mediche avanzate. Complessivamente siamo d'accordo con il testo a prima firma della collega Paita, ma riteniamo che debba essere chiesto con ancora più forza di assumere iniziative che contrastino il ricorso ai cosiddetti medici a gettone attraverso cooperative per i servizi ospedalieri che le aziende sanitarie locali non sono in grado di soddisfare, con particolare riferimento ai pronto soccorso. soccorso. L'uso distorto dell'esternalizzazione non soltanto genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta anche gravi criticità in termini di sicurezza, continuità e qualità delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia per la ridotta fidelizzazione di questi ultimi alle strutture pubbliche. La pandemia poteva essere l'opportunità per la politica di ripensare anche alcuni modelli. È quanto mai importante adottare tutte le iniziative di competenza perché la riorganizzazione della rete di medicina territoriale favorisca, attraverso l'azione congiunta delle diverse figure disciplinari e professionali medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, specialisti ambulatoriali, operatori sociali ed altro - un modello integrato che tenga conto non solo delle dimensioni di assistenza e cura prettamente medica, ma anche delle dimensioni sociali e contestuali della persona. Il definanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato particolarmente selettivo ed ha penalizzato principalmente il personale attraverso il blocco del *turnover* e dei contratti dei dipendenti, la dilatazione del lavoro precario e l'esternalizzazione dei servizi. Di tutto ciò hanno sofferto e soffrono sempre di più la qualità e la pronta disponibilità dei servizi per i cittadini, ai quali oltretutto è richiesto il pagamento di un'odiosa e spesso salata tassa di accesso ai servizi quale è diventata ormai il *ticket*, con due ordini di conseguenze: la rinuncia a curarsi per milioni di cittadini a causa delle troppo lunghe liste di attesa, dei costi eccessivi, della distanza dal luogo di cura, una rinuncia che ha colpito maggiormente - ma non solo i gruppi più poveri della popolazione e le Regioni meridionali; il ricorso sempre più frequente dei pazienti al settore privato in diretta e facile competizione col settore pubblico sia sui tempi di attesa, appunto, che sulle tariffe delle prestazioni. La tutela della salute di tutti - nessuno escluso - soprattutto dei più poveri, colleghe e colleghi, deve ritornare al centro delle nostre priorità e di quelle del Paese ed è per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.

I Gruppi hanno bisogno di leggere i testi delle riformulazioni e delle proposte di modifica avanzate, anche per poter tarare la propria dichiarazione di voto e l'indicazione di voto. Questo mi sembra essenziale cinque minuti sono sufficienti

io mi associo, anche perché il nostro Gruppo intende sostenere la mozione presentata e voterà favorevolmente. Colgo l'occasione anche per fare qualche considerazione. Prendo atto che anche questa volta il rappresentante del Governo precisa in maniera molto capillare che ci troviamo in una situazione che era stata prevista già in passato dal Governo precedente e questa è un po' una caratteristica di chi

da zero: ha preso in mano una nave che era in viaggio in mezzo ai marosi, a volte tempestosi a volte meno, che era stata portata fino a un certo punto da chi governava in passato e che verrà portata avanti da chi governerà in futuro. Il compito di chi governa ora è fronteggiare al meglio le problematiche e le circostanze del momento. In questo senso sento di associarmi *in toto* a quanto detto dalla senatrice Cucchi.

dai presentatori della mozione. Servono interventi strutturali e serve soprattutto che si stanzi denaro, ma in funzione di obiettivi chiari da raggiungere. Abbiamo problemi

propositiva. Ovviamente noi siamo a disposizione per ragionarci insieme, ma almeno fissiamo degli obiettivi che ci consentano di uscire dalla situazione estremamente critica

è indicativo dell'idea di Paese che si ha, delle sue priorità, dell'emergenza sociale che stiamo vivendo e anche di un approccio, visto che siamo spesso criticati anche per come conduciamo

tema dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese, che si manifesta anzitutto nel rischio che si metta in discussione un modello che prima veniva definito dalla mia collega Sbrollini come un modello di cui noi andiamo orgogliosi: l'universalità delle prestazioni, l'idea di una sanità pubblica che arrivi a dare risposta ad ogni cittadino.

Se non si riesce ad offrire una prestazione in tempi congrui, un cittadino che non si può permettere una prestazione di carattere privato ha due sole alternative: o fare i conti con questa emergenza e privarsi magari di altri bisogni altrettanto importanti per la propria vita, oppure rinunciare a curarsi. I dati dicono che purtroppo per moltissimi italiani la scelta obbligata è stata rinunciare a curarsi. Penso che non dovremmo avere altro assillo che questo, perché non c'è nulla di più ingiusto.

e hanno cercato di onorare il loro mandato in quella fase. Noi avevamo assunto come grande impegno collettivo il fatto di uscire da quella emergenza con un Sistema sanitario che fosse maggiormente in grado di dare risposte nei momenti di bisogno. Allora fatevi due conti: esiste davvero una quantità di posti in terapia intensiva maggiore rispetto a quando è scoppiato il Covid? Sfido chiunque a darmi dei dati che dimostrino che sono stati fatti dei passi in avanti. Esiste un miglioramento nelle liste d'attesa che sia in grado di dirci che oggi siamo capaci di prevenire e di dare risposte tempestive a chi ha bisogno di salute? Esiste una medicina territoriale che abbia saputo fare dei passi in avanti nel nostro Paese? No: tutto questo non è accaduto. è accaduto. Nessuno può gettare la croce addosso agli altri, perché qui c'è un problema strutturale complessivo che va ben oltre il mandato dei dieci mesi di questo Governo. Il nostro tentativo, però, è provare a lavorare tutti assieme, perché ci sia finalmente una risposta corale e un impegno di questo Parlamento nella direzione di una sanità che deve essere ripensata complessivamente, che il Sistema attuale non regge, e perché ci siano delle risorse che vadano a costituire un investimento duraturo e sistematico nei livelli sanitari territoriali, nelle diverse articolazioni e nelle diverse risposte che le Regioni danno. Se c'è un tema su cui io - lo dico con franchezza - non comprendo quale possa essere il beneficio dell'autonomia in questo Paese, è il tema della sanità. della sanità. *(Applausi)*. Vedere che ci sono Regioni nelle quali si è in grado di preventivare una risposta e Regioni nelle quali si è completamente abbandonati è qualcosa di inaccettabile. Ecco perché la discussione che facciamo ora si collega a quella che faremo dopo. Non ho ancora capito perché la faremo dopo e cosa sia successo nello stillicidio della maggioranza,

di compromettere complessivamente l'esigenza di salute del nostro territorio. Il Governo ci ha detto, seppur in modo sfumato, sfumato, che accetta le nostre proposte. Anche qui stiamo facendo un passo in avanti e io la ringrazio, signor Sottosegretario, perché solo pochi giorni fa abbiamo fatto un *question time* su questo punto e di risposte non ne sono arrivate. Oggi, anche grazie al fatto che noi ci siamo messi in gioco con una mozione

Diciamo però che lo prendiamo come un buon auspicio per continuare una discussione assieme. Nella legge di bilancio saremo in grado di vedere se è stato fatto o no qualcosa sul tema sanitario. Noi in piazza non dichiariamo di andarci prima della legge di bilancio: vediamo cosa ci scrivete e poi eventualmente valuteremo cosa siete in grado di fare per il Paese. la mozione ha evidenziato una serie di problematiche in ambito sanitario, ma si tratta di temi su cui il Governo e in particolare il ministro Schillaci stanno già lavorando e dando delle risposte concrete. Certamente i problemi della sanità italiana esistono, ma essa rappresenta ancora oggi uno dei modelli di tutela della salute in tutto il mondo. Io stesso, che vivo in una Regione del Sud, mi accorgo delle carenze del sistema sanitario campano, rispetto a quello di altre Regioni come la Lombardia o il Veneto. Ma so anche che nella mia stessa Campania esistono delle eccellenze che sono un modello per il resto del mondo. È però innegabile che i divari nelle prestazioni e soprattutto nei tempi di attesa devono essere affrontati in modo deciso, per dare risposte ai cittadini in lista di attesa. Si tratta di una dotazione strutturale che nel Mezzogiorno deve stare al passo con quella degli esempi più virtuosi. Ma c'è soprattutto un modello organizzativo della sanità pubblica che deve diventare omogeneo a livello nazionale. Quindi, c'è senza dubbio un tema da porre a livello nazionale, ma poi bisogna confrontarsi nelle sedi ulteriori dove la sanità viene gestita, che vedono dei confronti tra le diverse realtà regionali (da Agenas alla Conferenza Stato-Regioni), che adesso si confrontano con la grande sfida delle risorse del PNRR (Missione 6), che puntano a ridisegnare una sanità a livello territoriale. la sfida sta tutta nel portare a termine, oltre che le riforme, gli investimenti che puntano ad avvicinare la medicina ai pazienti. Crediamo che sia fondamentale il potenziamento dell'assistenza domiciliare anche grazie all'impegno della telemedicina. Seguiamo con interesse la realizzazione di nuove strutture e presidi sanitari sul territorio per migliorare l'accessibilità e ampliare la disponibilità dei servizi di prossimità ai cittadini. Quindi, vanno portati avanti i progetti che prevedono la creazione di 1.350 case di comunità per la presa in carico del paziente; così come quelli che vedono la creazione di 400 ospedali di comunità rinnovati, interconnessi e tecnologicamente avanzati; e ancora la realizzazione di 600 centrali operative territoriali per il coordinamento dei servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari (una ogni 100.000 abitanti), così come l'attivazione della telemedicina. Le risorse questa volta ci sono, posto che a questa finalità sono dedicate 7 miliardi di euro dal PNRR. Allo stesso modo, valutiamo positivamente il *focus* che si è fatto sulle Regioni meridionali. Nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia saranno investiti, attraverso il programma nazionale Equità nella salute, ulteriori 625 milioni di euro. Per queste Regioni è prevista l'attivazione di centri di prossimità contro la povertà sanitaria e azioni di educazione sanitaria. Rientrano tra i progetti anche il potenziamento dei dipartimenti di salute mentale e la promozione di interventi integrati in collaborazione con servizi sociali e terzo settore. previsti anche il rafforzamento e l'inserimento dei consultori familiari, il potenziamento dei centri regionali per percorsi di affermazione di genere e centri clinico-assistenziali rivolti alle persone transgender e di genere non conforme. Si prevede anche l'aumento della copertura degli *screening* oncologici. Questo intero programma è per le Regioni del Sud. ricordato infine che la Missione 6 del PNRR conta su 15,6 miliardi complessivi da investire anche in innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale: sono risorse che avranno certamente una ricaduta positiva se saranno utilizzate in modo puntuale. Molti dei problemi relativi alla carenza del personale medico e infermieristico che riguardano la loro remunerazione sono già stati affrontati da recenti provvedimenti del Governo.

noi crediamo che compilare un quaderno di lagnanze non serva a risolvere i problemi. Abbiamo la fortuna di avere un Ministro competente e determinato a portare avanti un nuovo modello di sanità pubblica e una maggioranza pronta a sostenere gli importanti impegni che lo aspettano. Annuncio pertanto il voto favorevole dei senatori di Forza Italia sugli impegni della mozione così come sono stati riformulati dal Governo. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

Generalmente la valutazione degli stanziamenti deve essere effettuata - ce lo dicono tutti gli studi di economia - in funzione al rapporto rispetto al PIL.

Sia personalmente, in qualità di senatore, che come rappresentante del mio Gruppo politico, non sono assolutamente favorevole alla richiesta di risorse provenienti dal MES.

puro ossigeno in realtà maschera di fatto una misura che rappresenterebbe soltanto un ulteriore debito sulle spalle di 60 milioni di cittadini. Come più volte abbiamo ribadito, i fondi stanziati dal PNRR andranno a potenziare il Sistema sanitario nazionale anche nella direzione prevista da questa mozione: pertanto, a nostro parere, non serve un nuovo prestito, un ulteriore macigno sui nostri giovani

Crediamo che, se non si fossero compiuti errori storici, come per esempio la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha decentrato la gestione della sanità, frammentando il Servizio sanitario nazionale in tante cabine di regia, oggi ci troveremmo in un'altra condizione. Siamo convinti, perciò, che migliorare la qualità media dei servizi ridurrebbe le disuguaglianze regionali, diminuendo i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche e per gli interventi terapeutici. Penso ai milioni di malati fragili italiani, spesso ammassati nei pronto soccorso, in attesa di ricevere le cure presso i poli ospedalieri. è positivo l'impegno volto a elaborare un piano pluriennale di interventi di prevenzione, così come lo è il richiamo nella riformulazione al piano di prevenzione. alla prevenzione anche in termini di prevenzione primaria: quanto è stato appostato in termini di prevenzione primaria? Il MoVimento 5 Stelle ritiene che la prevenzione primaria sia e debba essere uno dei pilastri della prevenzione. Condividiamo anche l'impegno volto ad assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale, applicando il sistema della medicina proattiva, rendendosi necessario il rinnovamento delle strutture ospedaliere, ovviamente trovando i capitoli di spesa adeguati, perché siamo ancora in attesa che il DM n. 77 dia i frutti delineati nel provvedimento.

debba essere un impegno specifico del Governo e richiamiamo per adesso la legge finanziaria n. 67 del 1988, *ex* articolo 20, che però non ha ancora consentito di mettere a terra i miliardi necessari per questo finanziamento. Onorevoli colleghi, ciò premesso, il MoVimento 5 Stelle

dovrebbero avere altri destinatari anziché il Governo, ma nell'interesse generale ce ne facciamo carico con la riformulazione di maggioranza. L'emergenza pandemica ha sottoposto il nostro sistema sanitario ad uno *stress test* che ci saremmo augurati, onestamente, di non dovere sperimentare mai. Altrettanto onestamente, al di là di talune indicazioni che possono considerarsi discutibili, ma che sarà giusto approfondire, il sistema nel suo complesso ha retto dignitosamente bene. È emerso che tali problematiche andranno superate e noi proponiamo soluzioni concrete, senza dimenticare la sostenibilità nel lungo periodo. Ecco perché una prima riflessione che si pone è quella di ricordarci che nessuno pensa che sia possibile superarle dall'oggi al domani, ma stiamo agendo affinché dieci anni di programmazione snaturante ed imprecisa non richiedano per porvi rimedio gli stessi tempi. Perciò, pur accelerando, sarà necessario almeno un quinquennio per arrivare ad un punto in cui le criticità evidenziate sembrino un brutto ricordo. Ci stiamo lavorando, in modo serio, pressante e condiviso, ma, a distanza di così poco tempo, pensare di vedere a terra i risultati è utopico. Difatti, solo per fare un esempio, la programmazione per le specializzazioni mediche, come tutti sapete, è un *iter* lunghissimo e noi di questo ci siamo occupati per il rilancio e il conseguente recupero di attrattività delle professioni mediche

dei contratti di formazione specialistica e per la valorizzazione dei contratti e dei ricercatori di alta specialità. Orbene, questa iniziativa legislativa è tale per cui ha sottesa l'intenzione di porvi rimedio in modo strutturale, così pure per quanto riguarda la carenza cronica di infermieri, ma, come dicevo, serve del tempo prima di vedere i risultati. Ciò a completamento di quanto puntualmente affrontato con i disegni di legge nn. 224 e 227, sia sul riordino dell'emergenza-urgenza, sia per il rafforzamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria, ordinamentali per il raggiungimento degli impegni assunti dal Governo nella risoluzione di accompagnamento al DEF approvata l'aprile scorso. È infatti evidente che i disegni di legge che vi ho citato andranno ad influire in modo significativo

di continuità assistenziale effettivamente integrato ospedale-territorio e adeguatamente upgradato in ammodernamento tecnologico e strutturale, per risposte più rapide e contemporaneamente più umanizzate verso i bisogni cronici e di bassa intensità, di primo livello e di primo intervento specialistico, in cui il medico di medicina generale

e all'implementazione di un sistema di valutazione delle *performance* degli erogatori molto attento alla prevenzione e all'appropriatezza. In conclusione, è nostro intendimento realizzare una strategia più ampia, che vada a coniugare l'incremento programmato delle risorse determinate e assegnate incidenti sul livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale in ragione dell'effettiva dinamica dei bisogni da tutelare e con la necessità di una riprogettazione complessiva del capitale umano dei professionisti della sanità, capace di contrastare sprechi e inappropriatezze, percorrendo una strada che dev'essere di oculata razionalizzazione, prima ancora di generare debito. Per tutto quanto appena detto, il nostro voto è perfettamente in linea con le riformulazioni analiticamente prospettate in maggioranza.

per rispondere all'intervento accorato del sottosegretario Gemmato. Signor Sottosegretario, il primo intervento di controllo della spesa, uno dei più importanti, più decisivi e forse anche più violenti nel Sistema sanitario nazionale è del 2007, efficace dal 2008, sul blocco del *turnover* del personale. la madre di tutti i problemi che abbiamo ad oggi ereditato. Sempre nel 2008 viene introdotto, per il controllo della spesa, il *payback* farmaceutico, da cui ancora oggi non riusciamo a uscire, sul controllo della spesa farmaceutica. Questi due eventi non non sono accaduti a caso, ma semplicemente perché, dopo la riforma del Titolo V del 2001, le Regioni erano quasi tutte commissariate e la spesa sanitaria non era più sostenibile. Dopo tali eventi, abbiamo avuto altre tre crisi: la crisi dei debiti sovrani,

di queste crisi strutturali del nostro Sistema sanitario italiano, del debito finanziario della salute, si è fatto carico praticamente l'intero arco costituzionale, nell'ultima fase, negli ultimi dieci anni, eccetto Fratelli d'Italia. Onorevoli colleghi, oggi anche voi siete al Governo e quindi, in questo momento, tocca a voi la gestione di questa fase. Tocca a voi, però con una novità: non c'è più la *spending review*; il patto di stabilità è sospeso; c'è il PNRR, con circa 20 miliardi di euro di finanziamento sulla parte degli investimenti; ci sono i fondi di coesione e sviluppo; c'è un piano dell'Europa completamente trasformato nella sensibilità sui temi della salute, basti pensare ai temi e alle risorse legate al cancro, con circa 4 miliardi di euro, come obiettivo e *goal* europeo. Quindi, oggi la situazione è fortunatamente cambiata. Voglio dire questo

grande come quella del Covid, da cui fortunatamente siamo usciti, ma di cui dobbiamo fare tesoro per poter riorganizzare la nostra programmazione sanitaria. Il 24 gennaio del prossimo anno si Il 24 gennaio del prossimo anno si incontreranno tutti i Ministri della salute in sede OCSE. Il tema, per i Paesi dell'OCSE, è come fare affinché i nostri sistemi sanitari reggano di fronte alle sfide enormi di salute pubblica che abbiamo dopo il Covid. La buona notizia è che "mal comune, mezzo gaudio". La cattiva notizia è che ci dobbiamo organizzare ed essere pronti a farlo.

persone anziane, con un'aspettativa di vita fortunatamente del più 7 per cento, ma con una domanda di salute, di bisogni pari a più 9,4 per cento rispetto a quello che noi spendiamo oggi. Il 2050 è domani e non tra cento anni. In questo contesto c'è bisogno di una presa di consapevolezza del Paese e dei decisori politici tutti, che deve cambiare musica sulla questione sanitaria. MEF, Ragioneria, guerre tra poveri; il Consiglio dei Ministri, prima di fare il bilancio, è un *suk*. Ma noi di quante risorse abbiamo effettivamente bisogno per fare le riforme che ci servono? La riforma del personale, non fare migrare il nostro capitale umano e le nostre eccellenze, riuscire a rendere attrattivo il nostro Sistema, pagare i debiti delle Regioni: tanto non c'è trippa per gatti finché quella partita non l'abbiamo finita. Che ci dicano che mancano 1,4 miliardi quest'anno, che ci dica il Ministro che ne mancano 3,3, finché la partita delle Regioni non è chiusa dal lato del bilancio, noi non riusciremo a garantire le prestazioni, cioè i LEA, le terapie ai ai nostri cittadini. *(Applausi)*. Quanto ci serve per riformare la prevenzione, evitare nuovi *virus*, nuove crisi, ma soprattutto passare dalla medicina di cura a quella che costruisce la buona salute, cioè proattiva, che fa della prevenzione, della medicina del territorio, di una riorganizzazione dei dei nostri sistemi territoriali, la barriera per dare risposte ai cittadini? Ci vogliono 7 miliardi. Sembrano tantissimi, ma non lo sono in quest'ottica, perché questi 7 miliardi garantiscono valore, economia, produttività, benessere e pace sociale per le nostre popolazioni. Troviamoli allora nella legge di bilancio, avviamo un percorso insieme. Non dico mica che vanno trovati tutti quest'anno, ma mettiamoli come una priorità.

Signor Presidente, colleghi senatori, sottosegretario Gemmato, la data di presentazione di questa mozione credo sia emblematica: 26 gennaio 2023. La voglio comparare alla data di insediamento di questo Parlamento e di questo Governo: ottobre 2022. in questa mozione c'è una elencazione di tante criticità e di tanti sfasci. Non possiamo credere che la causa e la responsabilità di tutto questo siano da addebitare a Fratelli d'Italia. *(Applausi)*. Possiamo anche condividere che oggi c'è un problema emergente, che è l'invecchiamento della popolazione, ma aggiungo l'emergere di patologie croniche degenerative è un problema non di oggi, ma anche di ieri, quando qualcuno che si è infervorato prima di me era il Ministro della sanità. Il sottosegretario Gemmato ci ha richiamato all'unità rispetto a questo tema. Ha detto che non dobbiamo dividerci perché la sanità non può essere né di destra né di sinistra. *(Commenti)*. A questo monito mi voglio anche

Tutte le questioni poste (il mancato potenziamento della prevenzione e della medicina territoriale e distrettuale, vetustà di strutture e di attrezzature, carenze di personale medico e infermieristico per mancata programmazione dei fabbisogni, liste di attesa, resistenza all'innovazione, perdita di attrattività delle professioni sanitarie) *(Applausi)* sono tutte derivate dal passato, noti al nostro Governo e al Ministero della salute e al ministro Schillaci, di cui ci stiamo facendo carico non perché

Il tema delle risorse diventa centrale e credo che il sottosegretario Gemmato abbia spiegato bene. Noi dobbiamo fare i conti tra una percentuale e l'ammontare del PIL, perché se si parla solo di PIL si dà un'informazione scorretta. Oggi, se dobbiamo essere veramente uniti, dobbiamo tifare affinché questo PIL cresca, affinché si dia credibilità al nostro Governo, affinché si dia sostenibilità al nostro Paese. Questo è quello che vogliamo e per questo confidiamo nell'azione del Governo Meloni. C'è un altro tema che dobbiamo affrontare,

in questo nostro Paese. Si è perso tanto tempo che noi vogliamo e dobbiamo recuperare, perché lo dobbiamo ai nostri elettori.

che il tema centrale è rappresentato dal reperimento delle risorse in questo nostro Paese e dalla crescita del PIL. Possiamo certamente, però, come Gruppo di Fratelli d'Italia, condividere il parere espresso dal sottosegretario Gemmato su tutti gli impegni che questo Governo assumerà, manterrà e porterà avanti. il voto del nostro Gruppo sarà conforme al parere espresso dal sottosegretario Gemmato in una relazione che ci rende orgogliosi, perché abbiamo ascoltato un impegno vero, serio, tecnicamente ineccepibile di un Governo che sta sul pezzo, che si pone sulle spalle i problemi e i bisogni di salute della nostra popolazione.

quali siano le materie riferibili a livelli essenziali delle prestazioni, quindi concernenti diritti civili e sociali, che saranno garantiti su tutto il territorio; in accompagnamento a tale subemendamento, il Governo produrrà anche le motivazioni che avranno portato

Senatore Borghi, non avvii malamente il suo incarico prestigioso.

La dichiarazione di voto è unica, non ci sono dichiarazioni separate sugli ordini del giorno. Allo stato noi abbiamo una richiesta del senatore Romeo, su cui l'Assemblea si deve pronunciare. Se sarà accolta, si potrà votare la mozione per parti separate, altrimenti no.

dice testualmente - e lo dico soprattutto ai colleghi della maggioranza, che hanno a cuore la trasparenza e la conoscenza dei dati e delle informazioni - che

la sede. BOCCIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, prima di votare quest'ordine del giorno - perché non ci è consentito intervenire - noi vogliamo capire se il Governo è contrario al trasferimento di dati e informazioni al Parlamento, non dei LEP, prima del voto

mi pare condivisibile. Peraltro il Ministro lo sa: questa richiesta di avere maggiori elementi di approfondimento sui LEP ci pare essere onestamente un atto dovuto. Avendo il Governo deciso di condizionare o comunque fortemente relazionare

purtroppo rimangono dei grandi non detti. Lo stiamo chiedendo da alcuni mesi, peraltro anche facendo riferimento a quanto è accaduto negli anni sulla sanità, dove sappiamo che esiste una sorta di equivalente dei LEP, ossia i livelli essenziali di assistenza (LEA), la cui determinazione non si è però tradotta, come purtroppo la storia di questo Paese dimostra in maniera inequivocabile, nel superamento delle diseguaglianze territoriali su un tema gigantesco come quello sanitario. Tanto è vero che, come sappiamo,

Questo nonostante i LEA, i livelli essenziali di assistenza, siano stati - quelli sì - determinati. Ora, dinanzi a questo punto, che a me pare però abbastanza inequivocabile, una risposta più chiara dal Governo la vogliamo e la chiediamo. Se questo è il tema di cui stiamo discutendo, ci basta davvero pensare che si possano semplicemente definire i LEP sulla carta, oppure bisogna necessariamente spiegare e capire, in primo luogo, come si finanziano i LEP dove si prendono i fondi per finanziarli e, in secondo luogo, il finanziamento dei LEP come affronta effettivamente il tema del divario territoriale? Altrimenti è evidente che anche i livelli essenziali di prestazione, così immaginati, rischiano di essere semplicemente un pannicello caldo e di non risolvere il tema di cui stiamo discutendo. È un tema serissimo e l'ho sottolineato anche quando ho cominciato il mio intervento

perché l'autonomia differenziata non c'è ancora, mentre invece i divari territoriali ci sono. Il punto è esattamente questo: se tale riforma diventerà effettivamente legge dello Stato, questi divari sono destinati ad essere ridotti o sono destinati ad essere accentuati? *(Applausi)*. Il timore è che questi divari siano destinati ad essere accentuati. Credo inoltre - ma qui siamo nel campo delle opinioni e ne discuteremo in altri momenti, anche quando avremo più tempo per argomentare - che, secondo me, sarebbe utile fare un lungo bilancio di questi vent'anni che ci siamo lasciati alle spalle. Lo dice uno che viene da una storia politica

«dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato», come se la Repubblica e lo Stato fossero due cose differenti *(Applausi)*, quando invece prima

completamente diversa e penso francamente che, dopo la pandemia e dopo quello che è successo in questi ultimi tre anni, nonché dopo i clamorosi fatti che hanno riguardato la sanità e che sono stati sotto gli occhi di tutti, insistere su questo terreno a me pare profondamente sbagliato. Spero davvero

una breve dichiarazione di voto, ricordando che l'articolo 5 della Costituzione sostanzialmente recita che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali e adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia. È in questo contesto che devono essere visti i provvedimenti relativi anche all'autonomia differenziata. Il testo proposto dal ministro Calderoli, sostanzialmente in attuazione del Titolo V, è quello Titolo V, è quello di una legge che determina la procedura e le regole, definendo successivamente le negoziazioni fra Stato e autonomie che chiederanno di esercitare l'autonomia differenziata. Come Gruppo non possiamo che essere favorevoli all'esercizio di funzioni e poteri a livello territoriale, ovviamente dentro un quadro normativo definito con legge dello Stato.

non parteciperà al voto su questa mozione, così come sugli ordini del giorno collegati e lo farà, non certo perché ritenga che la proposta di legge Calderoli sia da accogliere così com'è, al contrario, per ragioni di metodo oltre che di merito. Pur nel rispetto dell'iniziativa parlamentare di ogni singolo deputato e senatore, troviamo abbastanza singolare che, proprio nello stesso ramo del Parlamento nel quale in Commissione affari costituzionali si sta procedendo a un esame approfondito nel merito della legge, si voti questa mozione, non aiuti ad affrontare in maniera adeguata il provvedimento mentre in Commissione siamo in fase emendativa. esame è radicalmente contraria all'autonomia, che non lascia margine di manovra. Francamente non mi meraviglia, perché è la posizione che da sempre il MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno e trovo quindi che sia coerente con le posizioni espresse da sempre in questa materia. Un po' di sorpresa suscita semmai l'atteggiamento del PD, che all'inizio di questa legislatura ha presentato, non una, ma ben due proposte di legge sull'autonomia. Sorprende questo atteggiamento, ma prendiamo atto che evidentemente il vento dei 5 Stelle soffia forte anche in materia di autonomia. Ad ogni modo, crediamo nel lavoro che stiamo facendo vogliamo dire in maniera molto semplice quali sono i tre filoni emendativi che stiamo seguendo in Commissione. Innanzi tutto, come Azione-Italia Viva-RenewEurope, riteniamo fondamentale correggere il provvedimento di Calderoli, assegnando centralità e protagonismo al Parlamento, quindi ci sono emendamenti costruiti in questa direzione. Siamo molto, molto attenti e non ci accontentiamo di un ordine del giorno sul tema dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che sono il punto critico della proposta Calderoli. Non a caso, con Mara Carfagna ci siamo battute durante il Governo e ci siamo fatte interpreti delle esigenze del Mezzogiorno. Non a caso, abbiamo finanziato il LEP sugli asili nido: si tratta di 143.000 posti da attivare gradualmente, partendo da 120 milioni di euro iniziali previsti per il 2022, fino ad 1,1 miliardi a decorrere dal 2027. Proprio perché siamo attenti al tema dei LEP, pensiamo che non possa essere liquidato

maniera trasversale un pezzo della legge del Governo e non semplicemente un ordine del giorno. La terza questione riguarda le 23 materie del Titolo V: pensiamo per esempio che temi come l'istruzione e l'energia debbano restare fuori dall'autonomia. Su tutti questi aspetti noi ci siamo, ma riteniamo che il lavoro vada fatto in Commissione. Non è tempo di scontri ideologici, ma occorre fare passi avanti in concreto, votando gli emendamenti

che c'è un'invocazione da più parti sul fatto che l'autonomia sia graduale e bilanciata. Occorre fare in modo che non sia lo spacca-Italia, né lo scontro Nord-Sud, ma un elemento di cucitura e rammendo del Paese. Dovremo quindi avere la maturità di affrontare questo tema, favorendo il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni da Nord a Sud, ma intercettando i bisogni delle aree interne e depresse, della montagna delle piccole isole, garantendo la continuità territoriale. Se avremo la capacità di uscire dallo scontro ideologico e di perseguire un'autonomia bilanciata e graduale... *(Il ...avremo fatto l'interesse del Paese. Ecco perché Azione-Italia Viva-RenewEurope ha scelto di non partecipare al voto su una mozione che è fuori tempo, esattamente come gli ordini del giorno: in quest'Aula ne sono stati approvati tanti e francamente non hanno mai determinato grandi cambiamenti o grandi passi avanti per il Paese. Il lavoro va fatto in Commissione e lì sfidiamo il Governo a migliorare e, qualche volta, a cambiare profondamente la legge Calderoli. mi interrogavo su un assordante silenzio rispetto a questo disegno di legge e a questo progetto. Sono accadute infatti, in queste settimane, diverse cose, a partire dalla famosa relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che tanto scandalo ha destato ed è stata utilizzata un po' come una farsa anche dalla maggioranza per lanciarsi segnali interni l'un l'altro, come una sorta di pizzini, di allarmi reciproci; poi ci sono stati anche gli allarmi lanciati da organismi

Da ultimo ci sono state le dimissioni di quattro autorevoli componenti del comitato per i LEP, il CLEP. Mentre succedeva tutto questo, c'era una voce completamente assente: quella della presidente Meloni. Oggi, in quest'Aula, la presentazione di quell'ordine del giorno vergognoso svela il motivo del silenzio. Oggi la maggioranza si palesa e quindi anche la volontà della Presidente del Consiglio. In quest'Aula null'altro si sta svolgendo se non un mercimonio politico, un *do ut des* per per onorare il vecchio progetto della Lega Nord, oggi redivivo in un contesto sociale, politico, economico, sia nazionale che globale, completamente diverso da quando questo progetto fu fu concepito, negli anni Novanta. È un progetto che oggi stride ancor di più con la realtà in cui ci troviamo. Quindi oggi si spiega il silenzio della presidente Meloni. Qual è il punto? È uno scambio politico: l'autonomia differenziata, sostanzialmente il federalismo di fatto, il secessionismo di fatto,

Ha ragione la senatrice Gelmini: non ci sono soltanto il LEP, ma le criticità sono moltissime, a partire dal fatto che il Parlamento viene completamente esautorato, completamente escluso, anche a rischio di fare fare una legge anticostituzionale, perché invece, nel Titolo V, come modificato nel 2001, si prevede che tali accordi tra le Regioni passino per il Parlamento. Il Parlamento le vede invece soltanto di sfuggita, per dare eventualmente soltanto dei dei pareri non vincolanti. Onorevoli colleghi, se davvero si volesse lavorare in Commissione, come è stato suggerito, se davvero spirasse il vento del MoVimento 5 Stelle, cosa che sarebbe auspicabile, tutti qui dovremmo prendere atto di alcuni errori che sono stati commessi. È stato detto poc'anzi che il Titolo V è stato riscritto in maniera frettolosa, per andare incontro e cercare di sedare certi appetiti, sperando che potessero placarsi. Allora riscriviamolo, se non siamo i soli - e non siamo i soli - a temere che la cessione soprattutto di alcune competenze sia inattuabile sia inattuabile e impensabile, come per esempio quella sull'istruzione, o quella della tutela dell'ambiente. La tutela dell'ambiente! Ci rendiamo conto di cosa stiamo affrontando noi, oggi?

Se ci rendiamo conto di questo, dobbiamo anche capire che non è pensabile trasferire alle singole Regioni la tutela dell'ambiente e la protezione del territorio, cioè una strategia globale, non soltanto italiana, ma molto più ampia. la modifica del Titolo V, come chiede ad esempio il terzo impegno di questa mozione che andiamo a votare, è sì una cosa che si può fare in Commissione: si potrebbe fare tutto, davvero, per il bene del Paese. Il problema è che qui non siamo di fronte a un progetto per il bene del Paese, ma, come ho detto all'inizio, siamo di fronte a un *suk* istituzionale, a un mercimonio

Certamente condizioni di criticità in una riforma così complessa ci sono, le vediamo e le ha viste anche il Ministro che tra l'altro aveva anche approvato anche approvato alcuni di quei punti. È un contesto di innovazioni che sono necessarie per portare a compimento la riforma del Titolo V, che - vorrei ricordare -erano modifiche volute e approvate anche dalla sinistra. Come tutti i disegni di legge è un testo emendabile e quindi sarà l'esame della Commissione affari costituzionali a definirne la versione finale. Ci sono emendamenti e richieste anche da parte della minoranza, che vengono fuori da riflessioni costruttive a questi va prestata la giusta attenzione perché possono anche migliorare il provvedimento. E poi ci sono comportamenti meramente dilatori o di opposizione aprioristica al progetto, che tendono spesso ad inquinare il dibattito e ad ostacolare il percorso della riforma. Lo dimostra anche il fatto che non è stato voluto il voto parziale di questa mozione. di questa mozione. Forza Italia, in quanto forza liberale, rifugge da uno Stato centralista, che non sia fortemente ispirato al principio di sussidiarietà. Più si a problemi e alla responsabilità di chi governa, più facile ed efficiente può essere la soluzione a vantaggio dei cittadini. Del resto, anni di centralismo hanno concorso a creare o amplificare il divario e le diseguaglianze che ci sono in Italia.

politiche dirigiste, centraliste, tagli e trasferimenti da parte dello Stato agli enti locali che poi si riversavano anche nei LEP, nei servizi essenziali ai cittadini, il blocco del *turnover* che ha ridotto il numero delle persone disponibili anche di tecnici, di cui oggi paghiamo le conseguenze anche con l'applicazione del PNRR. E ancora pensiamo alla chiusura degli ospedali periferici

Ciò non toglie che la cautela per determinate aree ispiri in maniera predominante il nostro partito, che ha proposto correttivi a tutela del Sud e delle zone più svantaggiate del Paese attraverso emendamenti e ordini del giorno che sono stati da noi presentati. La questione meridionale per noi è nazionale, non solo per un principio di equità sociale rivolta a tutti i cittadini, ma perché l'Italia non può crescere se non si sviluppa il Mezzogiorno in modo sostenibile. Proprio per questi motivi abbiamo presentato ordini del giorno ed emendamenti ed emendamenti che tendono a riequilibrare i livelli delle prestazioni essenziali tra Sud e Nord, attenuando le condizioni di partenza. Secondo le nostre richieste qualsiasi intesa sottoscritta tra Stato e Regioni non deve pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna altra Regione, tenuto conto dei LEP. Inoltre, in un'ottica perequativa, abbiamo chiesto anche l'impegno del Governo a riequilibrare in prospettiva i LEP che riguardano tutte quelle materie oggi gestite a livello periferico, che già esistono. Questa riforma è certamente meno invasiva di quelle che in passato hanno già affidato ai territori l'85 per cento dei servizi. Parlo del trasporto pubblico locale e dei servizi sociali. È quindi essenziale prestare attenzione, non soltanto alle 23 materie che saranno soltanto alle 23 materie che saranno delegate con questa riforma, ma anche a quelle che sono già delegate come funzioni fondamentali agli enti territoriali. Al dato compensatorio

affinché alcuni servizi pubblici possano essere resi ai cittadini in modo più efficace e più efficiente di quanto non sia accaduto fino ad oggi. *(Applausi)*. Questo è l'unico obiettivo.

ministro Calderoli parla da sé e se ben letto, senza pregiudizi ideologici, risponde veramente a tutte le domande. Il regionalismo differenziato fa paura solo a chi non lo conosce o a chi non lo vuole conoscere.

che si potrà parlare di quali sono le risorse in relazione ad esempio ai singoli livelli essenziali quando sarà indicato quali sono i livelli essenziali e quando saranno quantificati i medesimi. Come si fa a sapere oggi se un domani sarà un livello essenziale il nucleo di valutazione multidimensionale di cui tratta una legge che ho sostenuto io quando sapremo quanti saranno i nuclei di valutazione multidimensionali, e se dovranno essere dei livelli essenziali. Se lo leggiamo attentamente, l'articolo 3 spiega come funziona il meccanismo economico e finanziario.

«I fabbisogni insieme alle capacità fiscali *standard* consentono, attraverso il meccanismo perequativo, di redistribuire con equità le risorse tra i diversi enti. In questo modo il meccanismo fondato su fabbisogni e capacità fiscali punta al superamento graduale del criterio fondato sulla spesa storica». Vi si dice, inoltre, che: fabbisogni e costi *standard* rappresentano un ecosistema istituzionale coeso e dinamico in cui esigenze diverse come efficienza e equità trovano una sintesi efficace e funzionale, capace di garantire tanto gli equilibri di finanza pubblica quanto i servizi necessari». Non stiamo parlando di qualcosa che non esiste, perché i LEP, i fabbisogni *standard*, i costi *standard* già ci sono nel nostro ordinamento e riguardano i Comuni,

Per questa ragione noi voteremo contro la mozione che è stata proposta, confermando ovviamente il voto a favore degli ordini del giorno della maggioranza con il parere favorevole del Governo.

è stata sottoscritta solo da forze politiche di opposizione, ma sarebbe importante che venisse sostenuta e votata all'unanimità e nella sua interezza, perché sarebbe un primo e significativo modo per dire ai cittadini, alle famiglie e alle imprese che si vuole ricondurre nei binari della Costituzione e dell'interesse generale l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e l'eventuale attribuzione a una o più Regioni di ulteriori condizioni e forme particolari di autonomia. Per quanto incerta e indeterminata possa apparire la formulazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è indubbio che tale disposizione non possa essere interpretata ed attuata in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, a partire dal principio di unità e indivisibilità della della Repubblica e al connesso principio di uguaglianza di fronte alla legge e nell'accesso a beni e servizi essenziali, che costituiscono l'oggetto dei diritti civili e sociali che, come esplicita appunto l'articolo 117, lettera devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Per garantire il rispetto di tali fondamentali principi, come è emerso anche nel corso delle audizioni e come abbiamo scritto nella mozione, mozione, prima di procedere a qualsiasi trasferimento di ulteriori competenze a una o più Regioni, occorre che siano determinati e concretamente attuati tutti i livelli essenziali delle prestazioni attinenti all'esercizio dei diritti civili e sociali. Colleghi, questo è un aspetto fondamentale molto importante, sul quale occorre da subito fare chiarezza. Come hanno spiegato anche Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Paino nella lettera con cui hanno motivato le loro dimissioni dal comitato per la determinazione dei LEP, se si procederà alla determinazione dei soli livelli essenziali relativi alle materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, vi è il rischio che alla fine manchino le risorse per finanziare i livelli essenziali delle prestazioni relativi alle materie di competenza esclusiva dello Stato. Pensiamo a materie come la previdenza sociale o, se preferite, a una materia come l'ordine pubblico e la sicurezza, di cui alla lettera *h)* dell'articolo 117 la predisposizione di un efficace presidio di forze di pubblica sicurezza, dotate di mezzi e di personale adeguati, non è forse l'oggetto di un diritto che deve essere garantito a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale? Con quali risorse pensiamo di garantirlo? Solo con quelle che residuano dopo che si è proceduto alla quantificazione e al finanziamento delle materie trasferibili alle Regioni? Come è di tutta evidenza, siccome le risorse sono necessariamente limitate e la definizione dello stesso concetto di essenzialità dipende dal loro ammontare, occorre che vengano determinati tutti i livelli essenziali delle prestazioni e che venga effettuata una valutazione complessiva delle risorse necessarie per finanziarli, superando ovviamente il criterio della spesa storica, che riflette e consolida diseguaglianze territoriali esistenti. Solo procedendo in questo modo il Parlamento sarà messo nella condizione di decidere priorità e grado della loro attuazione. Accanto alla predeterminazione di tutti i LEP, per ricondurre il confronto sull'autonomia differenziata entro i binari della Costituzione e dell'interesse generale, è poi necessario, come abbiamo scritto nella mozione, garantire un adeguato protagonismo del Parlamento nella determinazione dei LEP e dei contenuti dell'eventuale intesa. È poi necessario garantire la reversibilità di ogni processo di devoluzione e l'esclusione di alcune materie. Che senso avrebbe e quali e quanti danni produrrebbe, onorevoli colleghi, attribuire alla competenza esclusiva di alcune Regioni la disciplina, ad esempio, della produzione o della distribuzione nazionale dell'energia o delle grandi reti di trasporto e navigazione o del coordinamento della finanza pubblica o dell'istruzione o della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro? sgombriamo il campo da qualsiasi suggestione secessionista, da qualsiasi tentazione di dividere il Paese e di escludere alcuni territori dall'accesso a beni e servizi essenziali. Rassicuriamo il mondo dell'impresa, che in Commissione ci ha detto con chiarezza che le disuguaglianze, l'arretratezza strutturale e la povertà di alcune Regioni costituiscono un freno e una zavorra per l'intera economia e per le stesse Regioni più ricche e dinamiche. Votiamo a favore di questa mozione e poi trasformiamo il suo dispositivo in adeguate previsioni giuridicamente rilevanti. Concludo, onorevoli colleghi. Non rinunciamo a conoscere tutti i dati e tutte le valutazioni che ha fatto e sta facendo il CLEP. La conoscenza precede la volontà. Qualsiasi volontà libera e consapevole si può esprimere solo se conosce adeguatamente i dati di fatto presupposti. Come possiamo votare contro alla richiesta di acquisire tutte le valutazioni... *(Il microfono Concludo dicendo che non possiamo permetterci di rinunciare a richiedere al CLEP tutti i dati e tutte le valutazioni che ha compiuto e che sta effettuando.

per discutere al meglio questa mozione credo si debba fare una piccola digressione e tornare un po' al 2001, quando ci fu la riforma del Titolo V, una riforma per molti versi anche pasticciata, che però non ha voluto il Governo di centrodestra. Nella mozione, che è un po' anacronistica, sono riportate alcune doglianze da parte dei proponenti, tra cui anche le materie che sarebbero oggetto poi di delega alle Regioni. Alcune di quelle materie, ad esempio l'istruzione, non sono materie che il centrodestra ha inserito in quella riforma; l'avete voluta voi e oggi quindi vi lagnate di cose che provengono dalla vostra parte politica. *(Applausi)*. dell'autonomia differenziata forse potrà andare a colmare quelle lacune, con un confronto serio, che c'è stato. Devo ringraziare il ministro Calderoli e il mio presidente di Commissione, il presidente Balboni *(Applausi)*, perché grazie a loro si è aperto in Commissione un confronto davvero serio, che ha portato a fare oltre 50 audizioni, che ci hanno consentito di ascoltare in quella sede autorevoli giuristi,

audizioni, abbiamo avuto degli spunti. Tanto è vero che tutte le forze politiche hanno depositato degli emendamenti a questo disegno di legge, compresa Fratelli d'Italia. tutti emendamenti che cercano di migliorare, se necessario, il testo. In particolare mi riferisco a quelli del mio partito, che hanno tre capisaldi: rafforzare la coesione nazionale, ridare centralità o dare centralità al ruolo del Parlamento e soprattutto, quello che forse ci sta ancora più a cuore, aiutare le Regioni svantaggiate.

popolare e anche la fiducia che le Camere hanno dato al Governo, perché la fiducia si è basata su tutto il programma di Governo, che parla sia di autonomia differenziata che di nuove forme di elezione dei massimi vertici istituzionali. Ho sentito però parlare - e mi dispiace doverlo dire - per due volte in quest'Aula di mercimonio, una parola che sinceramente non avrei voluto ascoltare.

che si vuole aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e poi diventare essi stessi il tonno di quella scatoletta. Quello è mercimonio. *(Applausi)*. Noi procederemo rispettando il programma elettorale e i nostri impegni presi con gli italiani, garantiremo diritti civili e sociali agli italiani. Per questo annuncio che voteremo contro la mozione, salvo le parti per le quali c'è stato invece il benestare da parte del Governo e così sarà anche per l'ordine del giorno.

dei Gruppi di maggioranza saranno discusse in sedute successive in base all'andamento del calendario dei lavori, essendo poi prevista nel calendario la trattazione di argomenti non conclusi.

rappresentante del Governo, colleghi, prima di addentrarmi nell'illustrazione del testo della mozione, non posso per il tramite della Presidenza non ricordare al senatore Della Porta, che si lamentava di chi ha usato la parola mercimonio rispetto a quello che è accaduto sul testo della mozione e dell'ordine del giorno dell'autonomia differenziata, che la mia forza politica ha dovuto subire attacchi quando si è parlato di voto di scambio per il reddito di cittadinanza, che era nel nostro programma elettorale. *(Applausi)*. Si può non essere d'accordo sul reddito di cittadinanza poi forse il Paese vi farà cambiare idea - però ci avete accusato di voto di scambio che, anche nel lessico di questo Paese, credo che sia un po' più grave del mercimonio.

in evidenza e platealizza nel complesso ciò che per noi è evidente da tempo: Governo e maggioranza sono in totale confusione. C'è bisogno di un ordine del giorno al testo della mozione sull'autonomia differenziata per ricordare ai colleghi di Fratelli d'Italia che alla Lega del presidenzialismo non frega niente *(Applausi)* e a quelli della Lega da parte dei colleghi di Fratelli d'Italia che dell'autonomia differenziata non gliene frega niente. Abbiamo un Ministro che oggi dichiara che quello che sta succedendo al Nord e al Sud sono due facce della stessa medaglia - il cambiamento climatico - e la maggioranza presenta una mozione negazionista in cui dice che non serve fare niente: le industrie devono continuare a produrre come prima, perché tanto il cambiamento climatico è un'invenzione giornalistica. Viene accolta una mozione sulla sanità con il Sottosegretario che dichiara che il Governo sta investendo cifre astronomiche, quando è plateale il fatto che, invece, c'è una riduzione di un punto percentuale sul PIL degli investimenti in sanità e che la maggioranza e il Governo hanno intenzione di procedere procedere nel percorso di privatizzazione totale della sanità del nostro Paese. La proposta del MoVimento 5 Stelle, che è stata abbracciata dal Partito Democratico, da Alleanza Verdi e Sinistra, dal Gruppo è quella di istituire per legge un importo minimo orario lordo sotto il quale non c'è dignità per il lavoro. *(Applausi)*. È questo il punto centrale

il potere di acquisto dei nostri concittadini è diminuito in modo enorme e che solo nel nostro Paese si è avuto un calo del 2,9 per cento del salario medio annuale, laddove in Paesi che si prendono a modello di riferimento perché non hanno il salario minio - per esempio la Svezia Credo quindi che per la struttura del nostro Paese e delle politiche del lavoro del nostro Paese l'introduzione di un valore orario minimo sotto cui non scendere sia necessaria e questo non deve mettere in nessun modo in discussione la grande capacità di molti sindacati italiani e di molte forze sociali italiane che attraverso la contrattazione collettiva garantiscono i diritti ai lavoratori. È altrettanto evidente però che esistono ancora i contratti pirata e i contratti accettati e sottoscritti che invece prevedono tariffe orarie inferiori a quella che proponiamo noi: ad esempio, ricordo che stanno sotto quella cifra i contratti di servizi alla persona per il 67,1 per cento e i contratti di servizi alla ristorazione per il 44,6 per cento. Oggi il tema vero è consentire a chi lavora di avere uno stipendio dignitoso, che non umili il lavoratore *(Applausi)*: solo attraverso quella proposta riusciremo ad ottenere questo risultato. Concludo, signor Presidente, perché tra le varie discrasie di questa maggioranza ci sono un DEF che parla di moderazione salariale come elemento centrale per combattere l'inflazione e un ordine del giorno della maggioranza che dice che bisogna tutelare i redditi medio-bassi. Ecco, il Ministro dell'economia nel DEF scrive di moderazione salariale e l'ordine del giorno della maggioranza parla di tutela dei salari medio-bassi: mettetevi d'accordo; non so se state portando a sbattere questo Paese, perché non ho ancora capito dove volete portarlo.

da anni i salari si stanno riducendo, però la proposta del salario minimo, che abbiamo presentato unitariamente, ha aperto una discussione in questo Paese, volenti o nolenti, sul salario povero, il salario povero è determinato dalla precarietà, che ha prodotto l'abbassamento dei salari e ha indebolito la forza sindacale, l'unità dei lavoratori. Questo è il dato fondamentale. Siamo di fronte a questo dato.

che forse non sa di cosa parla. Non chiediamo assistenzialismo, ma chiediamo che i datori di lavoro paghino il giusto ai lavoratori e alle lavoratrici. *(Applausi)*. Questa è la cosa che bisogna fare.

anche con un contratto, prendono meno di 9 euro lordi. Credo che questo sia inaccettabile in un Paese civile. Concludendo, la nostra proposta non indebolisce la contrattazione. Vorrei rispondere al

Questo è il dato fondamentale ed è per questo che chiediamo di contribuire e di aiutare le aziende che arrivano a questo, perché la competizione si fa sulla qualità, non sui bassi salari e sulle condizioni di lavoro peggiori. La discussione che

una parte dei profitti ai salari e agli stipendi. Questa è la vera discussione in atto sul salario minimo.

Sono quasi 3 milioni i lavoratori e le lavoratrici che in Italia vivono sotto la soglia di povertà. Questo per un Paese civile non è accettabile. Il salario minimo esiste in quasi tutti i Paesi europei, compresi quelli che vantano tassi di occupazione e remunerazione ben più alti rispetto all'Italia. Ciò dimostra che non è un intervento che può alterare la dinamica tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, anche perché tale dinamica non è mai pura, ma ci sono interi settori in cui il lavoratore non ha alcuna possibilità negoziale nei confronti del datore di lavoro. Il salario minimo è uno strumento che quindi può creare un argine agli eccessivi squilibri e può contrastare quei rapporti di lavoro che rasentano lo sfruttamento. Si è detto in questi giorni che 9 euro lordi sono una cifra troppo alta. Invece ritengo che sia il minimo di civiltà. Se si pensa a quanto è aumentato il costo della vita, al modo con cui ciò impatta soprattutto sui lavoratori dipendenti al fatto che in Germania, per far fronte all'inflazione, a ottobre è stato portato da 9 a 12 euro l'ora. Non è un caso che questa proposta goda di un forte sostegno da parte dell'opinione pubblica. L'ultimo sondaggio pubblicato dai giornali di oggi dice che il 70 per cento degli italiani è favorevole, con punte importanti di consenso anche tra gli elettori di centrodestra. Sempre questo sondaggio dice che il 73 per cento degli italiani ritiene i 9 euro una cifra insufficiente e che una paga giusta sarebbe tra i 10 e i 12 euro l'ora. Insomma c'è una domanda che arriva dal Paese che non si può far finta di non vedere. È una domanda sul carovita, sul fatto che è inaccettabile lavorare ed essere una persona povera. Dire che un salario dignitoso sarebbe puro assistenzialismo è un atto di cinismo. Il Governo faccia un passo in avanti, ma lo faccia subito senza aspettare l'autunno. È con questo auspicio che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie alla mozione al

è dal 1990 che le retribuzioni medie lorde annue nel nostro Paese scontano un differenziale negativo e diverso rispetto ad altri Paesi con le nostre caratteristiche. Senza andare ad un confronto con altre realtà dell'Europa dell'Est o della Scandinavia e per rimanere al confronto con due Paesi che hanno le nostre dimensioni e le nostre caratteristiche, la Germania e la Francia, noi possiamo accorgerci che le retribuzioni medie in Germania dal Novanta ad oggi sono aumentate del 33,7 per cento, in Francia del 31,1 per cento e in Italia sono diminuite del 2,9 Se affianchiamo a questi dati la verifica sulla crescita in termini reali, che è passata dal 45 per cento del decennio degli anni per cento del decennio tra gli anni Dieci e gli anni Venti di questo secolo, cui è seguita la pandemia, ci rendiamo conto della complessità e dell'assurdità per alcuni aspetti. Vorrei però fare una domanda ai presentatori di questa mozione; esiste un nesso causale tra la mancata modernizzazione del Paese e la sua competitività? Esiste un nesso causale tra la debolezza della politica, la sperequazione dei redditi e il blocco dei salari? salari? Dopo un trentennio così, forse dovremmo riflettere sul fatto che la delegittimazione della politica, in cui molti si sono esercitati nel corso di questi anni, viene pagata dalle fasce più deboli della popolazione. E non basta, cari colleghi, per rifarsi una coscienza, una mozione degli affetti nei confronti dei più deboli. Bisogna riflettere sugli elementi strutturali che hanno intaccato nel profondo le istituzioni *(Applausi)*, impedendo loro di agire in termini di equità, di perequazione e di giustizia sociale. Cari colleghi del MoVimento 5 Stelle, tra questi elementi strutturali c'è stata anche l'azione sistematica di delegittimazione dei partiti, dei movimenti sociali e dei sindacati *(Applausi)* che solo recentemente state mettendo in discussione. Richiamo in proposito un interessante intervento del presidente Patuanelli sul «Corriere della Sera» di sabato scorso circa l'esigenza di ripristinare il finanziamento pubblico dei partiti. Forse vi state accorgendo anche voi che senza corpi intermedi, che con la piena disintermediazione, che con la rete al posto delle comunità, pagano i più deboli, paga un sistema di un mercato del lavoro che è sclerotizzato e che produce bassi tassi di occupazione, disoccupazione giovanile femminile, sacche di inattività. Evitiamo quindi per cortesia la logica settaria, secondo la quale chi è a favore del salario minimo è con i fragili e chi mostra delle perplessità è contro i deboli. Sappiamo bene infatti anche noi qual è il quadro e dobbiamo riflettere sugli strumenti. E se ci permettiamo di porre alcuni dubbi, lo facciamo esattamente per raggiungere lo stesso obiettivo. Diciamo, per esempio, di fare attenzione al rischio *boomerang*, all'abbassamento cioè della soglia delle retribuzioni sull'asticella fissata per legge, all'uscita dei contratti delle imprese che avrebbero una legge per diminuire la dinamica retributiva. Cari amici del MoVimento 5 Stelle raccontare che si risolve tutto con una legge ricorda troppo il balcone dell'abolizione della povertà e abbiamo visto come è andata a finire. Vuol dire non fare nulla? No. Abbiamo anche diverse sensibilità all'interno del nostro Gruppo e lavoreremo con le nostre sensibilità per raggiungere lo stesso obiettivo: politica dei redditi, taglio delle tasse sul lavoro, produttività a favore della crescita dei salari, sviluppo, partecipazione dei lavoratori agli utili. Non dimentichiamoci, cari colleghi, la lezione di Tarantelli, che lasciò la vita per queste cose. I salari si determinano in un confronto fra le parti sociali che tenga conto delle condizioni reali del mercato e la loro crescita è legata non all'inseguimento all'inseguimento dei prezzi al consumo, ma alla produttività, alla partecipazione dei lavoratori agli utili, alle concertazioni tra le parti sociali, in cui la politica svolge un ruolo di impulso ma non invade il campo. Se poi spiegassimo che dietro questa dietro questa proposta di salario orario lordo minimo a 9 euro c'è anche l'assorbimento comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive, delle indennità concettuali fisse e integrative, se spiegassimo che ci si propone di aumentare le tasse

che la politica si debba assumere delle responsabilità molto precise, non inseguendo la demagogia, non agitando in maniera generica delle bandiere e facendo annunci che poi rimangono tali, ma perseguendo una strada di autentica responsabilità. Come diceva qualcuno non dimenticato, la politica è altrove e prima o poi dovrete tornarci. Noi vi aspettiamo lì. Signor Presidente, «Se devi dire una bugia dilla grossa» è il titolo di una nota commedia che oggi la sinistra porta in Parlamento e nelle piazze per sostenere il salario minimo per legge. Di bugie, ma di quelle grosse, ne abbiamo sentite tante in questi giorni di campagna e di propaganda. Prima bugia:

lavoratori poveri, ci mancherebbe, ma aggiungendo che eventuali misure dovevano espletarsi nel rispetto delle competenze nazionali, quindi non c'è nessuna imposizione che arriva dall'Europa a fissare per legge un salario minimo orario. Al contrario, la Commissione riconosce che i Paesi con un'elevata copertura della contrattazione collettiva sono caratterizzati da un numero minore di lavoratori con stipendi bassi e con salari minimi sopra la media europea.

le sinistre - non si capisce se per amnesia o malafede - accusano il centrodestra di essere contro il salario minimo. Mi chiedo se sono le stesse sinistre che in questi anni hanno sfilato per strade e piazze, abbracciate con i sindacati come la CGIL che si sono strenuamente opposti a questa misura perché altrimenti avrebbero visto totalmente depotenziato, se non addirittura esautorato, il loro potere di contrattazione con le imprese. *(Applausi)*. Ci avete accusati sul punto di essere persino arroganti, ma vogliamo parlare dell'arroganza di chi, dopo aver governato per undici anni senza aver mai vinto le elezioni e pur essendo azionista importante, non ha mai avuto l'idea di proporre ciò per cui oggi dice di lottare e soltanto oggi fa proposte trabocchetto pensando di far fessi gli italiani? Terza bugia: il Governo e la maggioranza favorirebbero la proliferazione dei contratti cosiddetti pirata. Falso. Per dimostrarlo basterebbe leggere qualche libro di storia contemporanea, perché era il 1995 quando la sinistra politica e sindacale promosse uno sciagurato *referendum* sulla modifica dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. Fu questo *referendum* il padre di tutti i contratti pirata; da lì origina il fenomeno che vede pseudo-sindacati stipulare con organizzazioni di comodo, spesso molto poco rappresentative, accordi a danno dei lavoratori. Abbiamo tutti a cuore l'interesse dei cittadini, la dignità del lavoro e ovviamente stipendi adeguati, come infatti i provvedimenti del Governo hanno dimostrato. Sia ben chiaro, per evitare strumentalizzazioni, noi non siamo contro il salario minimo *tout court;* siamo contro la brutale semplificazione di un problema complesso. Imporlo per legge sarebbe controproducente e dannoso, perché in questo modo si rischia di spingere verso il basso anche i salari contrattuali presenti nella buona e sana contrattazione collettiva, che attualmente, come sappiamo tutti, sono più alti di 9 euro all'ora. modo volteremmo davvero le spalle ai lavoratori, perché guadagnerebbero di meno; inoltre si danneggerebbero i sindacati e la rappresentanza imprenditoriale, perché le aziende avrebbero maggior convenienza ad uscire dai contratti nazionali. Ci sono altri modi per aumentare i salari bassi, a cominciare dalla riduzione delle tasse e delle contribuzioni sul lavoro, cioè tagliando il cuneo fiscale e contributivo, come questo Governo sta già facendo. Infine vorrei sottolineare il rischio che la monopolizzazione del dibattito sul lavoro esclusivamente sul tema del salario minimo rischia di far cadere nel dimenticatoio il tema dell'adeguamento del salario complessivo, che è centrale. abbiamo annunciato la presentazione di una proposta di legge che ci auguriamo rappresenti finalmente la base di un dialogo senza ideologia, non tanto per introdurre una cifra oraria minima, ma per alzare le retribuzioni di di chi guadagna meno di 25.000 euro lordi. Tale proposta ha diversi obiettivi: continuare sul solco già tracciato della detassazione della tredicesima mensilità, del lavoro notturno e degli straordinari ed estendere ad ogni forma di assunzione la contrattazione collettiva già in essere fra sindacati e datore di lavoro, che già prevede livelli minimi di retribuzione. In questo modo combatteremmo lo sfruttamento del lavoro, il *dumping* e il lavoro sommerso. Per questi motivi non possiamo votare a favore della mozione n. 8. In conclusione, colleghi, se avete davvero a cuore il futuro dei lavoratori, smettetela con inutili ribalte e sedetevi a confrontarvi nel merito, altrimenti vorrà dire che la vostra priorità non è mettere più soldi nelle loro buste paga, ma strumentalizzare i bisogni e le sofferenze per lucrare qualche zero virgola nei sondaggi, ma non ci riuscirete perché non smetteremo mai di smascherare le vostre bugie e le vostre false soluzioni. Signora Presidente, sono un po' in imbarazzo dopo le affermazioni della collega che mi ha preceduto che, in quanto a bugie e travisazioni della realtà, credo abbia fatto il doppio salto mortale carpiato quest'oggi in Aula.

con meno di 25.000 euro di reddito annuo. Facendo due conti, se quei lavoratori fossero 3,5 milioni (ed è matematica spiccia che si impara alle elementari), avrebbero

l'anno sono ben più di 3,5 milioni, per cui sarebbero ancora meno dei 285 euro l'anno di cui ho parlato io, che equivalgono a circa 25 euro al mese. Ridicolo: questo è l'unico termine che si può dare a questa proposta *(Applausi)*. Se volete parlarne seriamente, facciamolo con delle proposte adeguate e metteteci i soldi, che però non andrebbero presi dalle tasse e dalla detassazione, perché quei soldi servono per dare servizi ai cittadini. Invece, l'aumento di stipendio dovrebbero pagarlo quegli stessi imprenditori che fanno miliardi di extra profitti; invece vogliamo tagliare i fondi statali e la contribuzione, contribuzione, quindi togliere altri servizi ai cittadini italiani. Così direi che non ci siamo proprio. Riprendo da quello che doveva essere il mio intervento in dichiarazione di voto. L'articolo 36 della Costituzione l'abbiamo imparato tutti, perché ho visto che viene citato anche nell'ordine del giorno della maggioranza, ma mi piace leggerlo: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Bene, gli articoli di giornale degli ultimi mesi recitano: «Salario minimo, sentenza del tribunale di Milano: pagare 3,86 euro all'ora è contro la Costituzione» (6 aprile). «Salario minimo: pagare troppo poco è anticostituzionale» (2 maggio). Arriviamo al 18 luglio: «Sfruttamento dei lavoratori, una nota azienda di vigilanza sottoposta a controllo giudiziario», perché pagava troppo poco, faceva caporalato e sfruttava i lavoratori. Quindi di sicuro un problema ce l'abbiamo. Uno dei comparti maggiormente colpiti dalla piaga delle paghe troppo basse è il contratto della vigilanza e multiservizi, che hanno un contratto collettivo, oltre ad averne di privati, ma anche quello sottoscritto dalle firme più rappresentative dei sindacati sta sotto i 9 euro l'ora (viaggia intorno a 6,50 euro per la vigilanza armata e a meno ancora per quella non armata). La stessa cosa per il personale che lavora nelle RSA, intorno ai 6 euro l'ora, come ha dichiarato più volte la mia collega Guidolin. Ci sono esimi costituzionalisti che dichiarano che il salario minimo deve essere stabilito per legge, visto che già lo fissava in origine la Costituzione. Sono un paio di giorni che la maggioranza comincia ad aver capito questo discorso, tant'è che oggi hanno avanzato una loro proposta e pensano di discuterne alla Camera, cercando di rinviare il voto sul disegno di legge delle opposizioni, perché c'è un sondaggio che dice che più del 70 per cento degli italiani è a favore, compreso chi sostiene il Governo. E finiamola anche con la barzelletta che il salario minimo a 9 euro l'ora porterebbe al ribasso gli stipendi che attualmente sono più alti, perché, se quello è il livello minimo, automaticamente deve essere riparametrato tutto verso l'alto ed è a questo che serve la contrattazione sindacale, è in questa direzione che va assolutamente rafforzata. Non dimentichiamoci di quello che ci chiedono i giovani, visto che parliamo continuamente di fuga dei cervelli che i nostri giovani se ne vanno all'estero. La loro di richiesta è di avere salari adeguati al costo della vita. Negli anni Ottanta con lo stipendio medio di un operaio si potevano comprare 1.000 coni gelato; fatte le dovute proporzioni, al giorno d'oggi non se ne acquistano neanche 500. Fatevi una domanda, rendetevi conto delle condizioni in cui vivono i lavoratori italiani e di quanto potere d'acquisto hanno perso. Gli altri 21 Paesi europei, che hanno già un salario minimo introdotto per legge, non hanno visto la contrattazione collettiva ridotta, né sono stati rivisti al ribasso gli altri salari. Ma naturalmente noi siamo sempre migliori degli altri e gli altri sono sempre degli sciocchi. Con la nostra proposta non sarebbero 280 scarsi gli euro in più all'anno nelle tasche dei lavoratori, perché 3,6 milioni di lavoratori che oggi guadagnano meno di 9 euro vedrebbero aumenti medi che partono da circa 800 euro. Questa è una proposta concreta per aiutare i cittadini italiani che sono più in difficoltà, i *working poors*, quelli a cui avete tolto anche l'integrazione del reddito di cittadinanza. È per queste ragioni che voteremo a favore della nostra mozione. *(Applausi)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe senatrici e colleghi senatori, sottosegretario Durigon, sono mesi che viene portata avanti una strumentalizzazione vergognosa da parte delle opposizioni,

di legge sul salario minimo: una del PD e una del MoVimento 5 Stelle. Nel Governo Conte 2, il Ministro del lavoro era dei 5 Stelle, mentre nel Governo Draghi il ministro del lavoro era Orlando. Allora mi chiedo: non ci credevate nemmeno voi o servivano solamente per strumentalizzare la questione? Partiamo dall'ABC. La questione si è naturalmente evoluta dopo l'approvazione della direttiva europea del 14 novembre 2022. Lo dice la stessa parola, "direttiva europea": dà indicazioni ed è una normativa che deve essere applicata a livello nazionale. La direttiva forse qualcuno non l'ha letta, non fissa una soglia europea del salario minimo, bensì detta le regole dentro le quali ciascun Stato membro deve muoversi. L'obiettivo dell'Europa non è quello di uniformare i sistemi nazionali sui salari minimi per la definizione di un salario minimo unico per tutti gli Stati membri europei, ma piuttosto di tendere direttamente a una convergenza

fine della direttiva europea, che però non si raggiunge. Il nostro Paese gode di una contrattualizzazione collettiva che copre l'85 per cento dei lavoratori. Questo sistema garantisce una serie di misure che negli anni sono state introdotte a tutela dei lavoratori: oltre al minimo tabellare c'è il TFR e la tredicesima, ci sono le ferie e i permessi. Tale sistema già in molti casi determina salari molto più alti del salario minimo. Le principali voci contro l'introduzione del salario minimo legale non provengono dalla Lega o dal centrodestra, ma direttamente dai sindacati dei lavoratori

descritto in precedenza. È vero, ci sono contratti i cui importi andrebbero aggiornati: mi riferisco a quello dei metronotte, la vigilanza armata o non armata, il cui salario è sicuramente inferiore al salario quello delle badanti, degli OSS all'interno delle RSA, delle *baby sitter*, delle *tagesmutter* che lavorano per le cooperative. Per non parlare poi delle notizie di stampa, dove si parla di cooperative che sfruttano i lavoratori immigrati all'interno del settore dell'agricoltura,

Altro discorso sono i contratti pirata: si tratta, come è noto, di accordi sottoscritti da organizzazioni sindacali per lo più fittizi, di comodo o comunque sprovvisti di adeguata rappresentanza sul piano nazionale. nostra Costituzione si tutela il lavoratore, secondo l'articolo 36, ma poi l'articolo 39 non è mai stato attuato. Allora è questo discorso che dobbiamo andare ad analizzare. L'introduzione del salario minimo metterebbe a rischio il sistema della contrattazione collettiva con il serio pericolo di favorire la tendenza alla diminuzione delle ore lavorate, l'aumento del lavoro nero, l'incremento della disoccupazione e l'aumento dei contratti di lavoro irregolari e dei contratti pirata. Addirittura potrebbe avere un effetto inflazionistico, a discapito dei salari che già superano la soglia del salario minimo. Una domanda importante riguarda il tema del lavoro e dei contratti, che non è sicuramente semplice. Come dicevo prima, c'è il *dumping* fiscale e il *dumping* salariale che va considerato a livello europeo. Con questo, non sono a dire che nel nostro Paese la contrattazione collettiva è perfetta; anzi, alla Camera è stata approvata una mozione in merito a novembre ed è in discussione il disegno di legge sul salario minimo. Nella mozione di maggioranza è stato votato il necessario rafforzamento della contrattazione collettiva, in linea con la direttiva europea, per estendere l'efficacia dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi anche in quei settori in cui effettivamente non ci sono. Vi è poi l'impegno a contrastare i cosiddetti contratti pirata da parte delle cooperative spurie, con particolare riguardo alla contrattazione di secondo livello e ai cosiddetti contratti di prossimità o ai contratti di distacco. Infine vi è un tavolo di confronto finalizzato alle politiche per la riduzione del costo del lavoro e all'abbattimento del cuneo fiscale: altro tema molto importante

per la dignità delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori. A proposito di questa battaglia - che oggi si consuma, non soltanto qui, ma poco lontano da noi a Montecitorio da noi a Montecitorio - ringrazio i colleghi del MoVimento 5 Stelle per avere voluto presentare una mozione su questo tema. In questa mozione riconosciamo i nostri obiettivi e i nostri valori, ma soprattutto qui sta l'ambizione di dare finalmente attuazione all'articolo 36 della Costituzione, che indica al legislatore la necessità, anzi, vorrei dire il dovere di riconoscere una giusta retribuzione al lavoratore, una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro,

libera da ogni ricatto e dignitosa in ogni sua parte. Al riguardo sarei davvero curiosa - ho ascoltato alcuni interventi - di approfondire realmente e di sentire argomentazioni su come si pensa di poter, non dico raggiungere, ma avvicinare almeno l'obiettivo indicato dalla Costituzione restando al di sotto dei 9 euro all'ora. all'ora. Stiamo parlando di 9 euro all'ora e credo che ognuno in quest'Aula dovrebbe mettersi davvero la mano sulla coscienza prima di aprire la bocca a casaccio, sparando parole in libertà, quando parliamo di 9 euro all'ora per il salario minimo: 9 euro lordi all'ora. *(Applausi)*. Comprendo l'imbarazzo della maggioranza,

si spiega non essere esattamente quello che si voleva ed è un'altra cosa. Ma l'imbarazzo che la maggioranza prova di fronte a tutto questo è tradito dall'ordine del giorno che è stato presentato oggi in quest'Aula, un ordine del giorno che è tutto benaltrismo: bisogna fare di più e meglio, ma l'importante è non fare ciò che è possibile, cioè votare insieme il salario minimo. e credo che dobbiamo riflettere un attimo e provare a ripercorrerli, invece che liquidare il tema, facendo ricorso all'argomento che ho appena sentito della contrattazione sindacale e dei contratti siglati siglati dalle organizzazioni sindacali. Parliamo di circa 3 milioni di lavoratori dipendenti, l'11,7 per cento di lavoratori dipendenti che riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali. Si tratta di una percentuale ben al di sopra della media europea, che si attesta al 9,6 per cento, altro che *dumping* salariale: *dumping* salariale: sono oltre 2,5 milioni i lavoratori che percepiscono retribuzioni al di sotto. L'insufficienza dei salari percepiti dai lavoratori italiani risulta confermata da un dato INPS che dovrebbe davvero colpire tutti noi che siamo qui a rappresentare il popolo italiano. Il dato INPS ci dice che l'insufficienza dei salari è tale che 365.000 persone titolari di un rapporto di lavoro attivo percepiscono in realtà il reddito di cittadinanza, che con il decreto-legge che avete votato ci apprestiamo a cancellare. Significa che sono lavoratori che percepiscono stipendi che non consentono loro di superare la soglia di povertà. Quando avanziamo la proposta di salario minimo, la cui soglia a tutela della dignità, come ho detto, è fissata a 9 euro, non parliamo del trattamento economico complessivo (anche questa è una cosa sbagliata che ho sentito pronunciare poco fa), ma di quello minimo. Emerge dai dati pubblicati in più sedi e vorrei citare semplicemente il «Sole 24 Ore», organo d'informazione della Confindustria: da una serie di importanti contratti collettivi nazionali, firmati dalle più rappresentative organizzazioni sindacali e datoriali, emerge che il parametro dei 9 euro orari non è rispettato in sei dei dodici profili professionali indicati. Sono numeri che sono stati pubblicati pubblicati l'8 luglio scorso, non farete fatica ad andarli a consultare. Sono stati citati alcuni dei profili e dei lavori nei quali si scende molto al di sotto dei 9 euro, come la logistica:

ebbene, i *rider* in bici non guadagnano neanche 9 euro lordi l'ora, ma sono fermi a 8,86. L'imballatore nella distribuzione moderna è

al di là della propria appartenenza politica, questo tema, che ha a che fare con la dignità della vita delle persone. Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

da quello che si è lasciato trasparire in questi giorni con le tante polemiche. Fratelli d'Italia e il centrodestra non hanno mai detto una sola volta che non ci sono salari troppo bassi. Non l'ha mai affermato, non l'abbiamo mai detto.

ci avete messo anni a capire che la Costituzione parla di una retribuzione che sia coerente con il lavoro fatto, perché, se ci aveste messo meno anni a capirlo, forse avreste fatto proposte precedenti e le avreste già approvate. E adesso dite a noi rinfacciate di non sapere che in Italia ci sono lavoratrici e lavoratori che guadagnano troppo poco? Lo dite a noi, che come prima mossa economica, già nella legge di bilancio, abbiamo tagliato il cuneo fiscale per dare soldi in più a chi guadagnava poco, cosa che voi non avete mai fatto in tanti anni di Governo? Voi dite questo a noi, rinfacciandoci che non lo sappiamo o che diciamo esattamente il contrario? No, la vostra è solo propaganda, è solo propaganda, per riavvicinarvi a quei lavoratori di cui per troppi anni non avete parlato e vi siete dimenticati. E adesso, prima dell'estate, parlate di salario minimo? Adesso?

come dire, va incontro alle esigenze dei poveri o di chi lavora poco e chi non lo è: non è così, signori, perché anche noi abbiamo presente cosa bisogna fare.

A chi mettiamo a carico quei 6,5 miliardi di euro? Al pubblico? *(Applausi)*. Non penso, perché lo stesso Cottarelli, che fino a poche settimane fa è stato senatore del del Partito Democratico, oggi ha detto che non si può pensare di metterlo a carico del pubblico. Allora lo mettiamo a carico del privato? Mettendolo a carico del privato, quante aziende sarebbero costrette a chiudere o a licenziare? Quanti posti di lavoro metteremmo a rischio con questa misura? Vi faccio l'esempio di una badante, delle tante badanti il cui stipendio contrattuale è di 7,80 euro all'ora. Una badante, messa in regola per trentotto ore a settimana, guadagna netti, in busta paga, 1.440 euro al mese.

ha detto che non è possibile il salario minimo come l'avete previsto voi, che il salario minimo deve essere quello stabilito contrattualmente per le varie categorie. Allora vedete che, se anche voi siete d'accordo a risolvere il problema,

questo problema, che noi non neghiamo. Onorevoli colleghi, vi invito a ritirare la mozione in esame, a non andare a uno scontro che non serve a niente e a nessuno, neanche a risolvere il problema. Serve solo a mettersi una medaglia nel mese di agosto, per poi tornare a settembre con lo stesso identico problema. Ritirate questa mozione, altrimenti il nostro voto sarà negativo, perché la mozione non serve a niente, non dice dove trovare i soldi, né come trovarli, se non, come qualcuno ha detto - questo è veramente incredibile - togliendo una parte del profitto a quelle poche aziende che ce l'hanno, per trasmetterlo ai lavoratori. Ciò significherebbe condannare a morte tantissime aziende, non tutte, non quelle che fanno extraprofitti, ma tantissime aziende che in questi momenti di crisi

Signor Presidente, colleghe e colleghi vorrei anzitutto ringraziare il collega Mirabelli *(Applausi)*, primo firmatario di questa mozione,

di politiche abitative nei miei dieci anni da assessore a Pisa; prima con la delega alle case popolari e nei successivi cinque anni anche come assessore all'urbanistica, imparando che su questi temi serve una grande capacità di ascolto e di visione. Tutto ciò che decidiamo di fare oggi non ha infatti solo una conseguenza nell'immediato, ma può cambiare i destini di migliaia di persone, il tessuto sociale di un quartiere e di una intera città. Quella che stiamo discutendo è una mozione che impegna il Governo su diversi punti. Su alcuni di essi, come è del tutto evidente, vi chiediamo un cambio di rotta. Nella scorsa legislatura infatti era stato rafforzato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, con un incremento di risorse di 160 milioni di euro per il 2020 e altrettanti per il 2021, oltre all'incremento per il Fondo morosità incolpevole. Con la legge di bilancio del 2023 queste risorse sono state spazzate via del tutto. *(Applausi)*. Ecco, io penso che chiunque abbia fatto l'assessore alla casa, (a chi tra i colleghi di maggioranza non è capitato di fare questa esperienza, rivolgo l'invito a fare una telefonata ai propri amministratori per poter verificare quello che sto dicendo). sto dicendo). Sappia che queste risorse servono a migliaia di famiglie italiane per non farle cadere in uno stato di povertà *(Applausi)*, per non costringerle a vivere una situazione di sfratto.

un segnale forte e importante verso cittadini che hanno bisogno di sentire il sostegno delle istituzioni *(Applausi)* e ne hanno bisogno ancor di più in una fase come quella che stiamo vivendo, nella quale l'aumento dei prezzi, l'inflazione che mangia i salari e le grandi difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro stanno acuendo sempre di più le già profonde diseguaglianze. È per questo che nei punti di questa mozione chiediamo al Governo un impegno più largo, come dicevo prima, un'azione che abbia una visione lunga e che vada incontro anche ai tantissimi giovani che si ritrovano ad affrontare, tra le tante difficoltà, quella dell'acquisto o dell'affitto di un immobile, oppure quella di trovare un alloggio ad un costo sostenibile nella città nella quale studiano. Nella società che stiamo costruendo, da una parte, c'è chi riesce, per patrimonio o liquidità accumulata, ad accedere al credito e all'acquisto di una casa, dall'altra, e sono soprattutto i giovani, chi non riesce a fare nessuna delle due, oppure chi riesce a farlo, ma con grande difficoltà e grazie al grazie al sostegno dei propri genitori e, ancora, alle esigenze di chi è costretto ad osservare inerme l'aumento dei tassi di interesse sui mutui che stanno letteralmente mettendo in ginocchio intere famiglie. Su questi aspetti chiediamo al Governo di intervenire anche nell'ottica della tanto sbandierata

per incrementare significativamente l'offerta di alloggi a canone sociale. Accanto a questo - è un punto che mi sta particolarmente a cuore - c'è la riqualificazione degli edifici pubblici sfitti per mancanza di manutenzioni straordinarie. È un tema di giustizia sociale: come possiamo accettare l'idea che ci siano tante famiglie che aspettano da anni l'assegnazione di una casa popolare sapendo che ci sono case sfitte che i Comuni non possono assegnare perché non hanno le risorse per manutenerle o rimetterle a posto? Di fronte a un'ingiustizia così evidente non possiamo girarci dall'altro lato. Il PNRR da questo punto di vista può e deve essere la grande occasione da sfruttare e anche su questo chiediamo al Governo un impegno concreto, immediato, fattivo e di lunga durata su un tema che può cambiare e migliorare la vita di milioni di cittadini italiani. La parola "casa" porta e deve portare con sé sentimenti positivi, finché per qualcuno rappresenterà sentimenti di ansia, paura e preoccupazione, nessuno di noi potrà sentirsi con la coscienza a posto.

Signor Presidente, nel ringraziare per l'opportunità di discutere del tema e ovviamente interessato al dibattito che si svolgerà in Aula e a cui evidentemente presterà grande attenzione relativamente agli orientamenti di voto che i Gruppi intenderanno esprimere,

sul secondo impegno il parere è favorevole subordinatamente alle seguenti modifiche, ovvero: inserire in *incipit* le parole «compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica», che è una formula che, come i colleghi sanno bene, accompagna inevitabilmente gli atti di natura parlamentare rispetto a ciò che non è nella programmazione; le parole «una legge quadro», inoltre, verrebbero sostituite dalle parole «un piano», evidentemente con ciò deflettendo dall'ipotesi di un intervento di natura legislativa. Sul terzo impegno il parere è favorevole subordinatamente alla seguente modifica: le parole «ottenere il saldo zero del consumo del suolo» sono sostituite dalle parole «ridurre il consumo del suolo», questo anche in ragione del fatto che, come i colleghi sanno, la materia è disciplinata da una concorrenza legislativa con le Regioni e pertanto si introdurrebbe un principio di facile censurabilità in sede costituzionale. Sul quarto e sul quinto impegno il parere è favorevole. Sul sesto impegno il parere è favorevole subordinatamente alle seguenti modifiche: sono inserite in *incipit* le parole «a valutare l'opportunità di»,

il parere è favorevole subordinatamente alle seguenti modifiche: le parole da «una più efficace» fino a «urbanistica delle città» sarebbero sostituite dalle parole «la revisione della disciplina delle locazioni di tipo turistico», quindi evidentemente eliminando una edulcorazione che ha più una connotazione di merito. Sull'ottavo, sul nono e sul decimo impegno il parere è contrario. Sull'undicesimo impegno il parere è favorevole subordinatamente alla seguente modifica: le parole «a utilizzare» sono sostituite dalle parole «a valutare l'opportunità di utilizzare», mentre il resto dell'impegno rimane immutato.

le parole da «a monitorare» fino a «incentivi fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare iniziative di competenza volte a rivedere le agevolazioni fiscali sulla casa e i *bonus* sul recupero edilizio e l'efficienza energetica».

«riportando l'agevolazione maggiormente nell'alveo della necessità di ammodernamento, efficientamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente,». Sul quattordicesimo impegno il parere è favorevole, così come sul quindicesimo, ma con le seguenti modifiche: le parole «ad adottare» sono sostituite dalle seguenti: «a valutare la possibilità di adottare»; le parole da «con allungamento» fino a «mutuatario» sono sostituite da: «anche eventualmente concordando con le banche forme di allungamento della durata

immutato. Sul diciassettesimo impegno il parere è favorevole subordinatamente all'accoglimento della soppressione delle parole da «prevedendo» fino a «rimborso del mutuo». Sul diciottesimo punto il è parere favorevole limitatamente alla prima

una cifra distintiva, quindi la vorremmo mantenere. Per tutte queste ragioni, noi non accettiamo

di cui circa mezzo milione sono minori - il che significa non potersi permettere le spese minime per condurre una vita dignitosa. Secondo poi i dati de «Il Sole 24 Ore», gli sfratti eseguibili in Italia erano circa 150.000, A questo proposito vorrei sottolineare che è stato addirittura azzerato il fondo contro la morosità incolpevole: siamo di fronte a questo dato.

maggiormente in difficoltà è quello di persone anziane per alcuni versi, di uomini e donne separate con figli, di giovani adulti che hanno un lavoro precario o disoccupati da molto tempo, perché la mancanza di lavoro e i bassi salari, di cui abbiamo discusso prima, portano ovviamente alla difficoltà di decidere tra il pranzo e la cena o l'affitto: si tratta quindi di una morosità incolpevole.

porre il problema di avere affitti abbordabili: molto spesso si tratta di giovani provenienti da famiglie composte da lavoratori e lavoratrici, impiegati, gente che lavora, che però non possono permettersi il caro affitti che c'è nelle grandi città universitarie,

oggi i mutui sono insostenibili; i mutui a tasso fisso sono passati da 300-400 euro a 800-900 e ci sono persone che devono decidere come mettere insieme il pranzo e la cena. La domanda è se se intendete intervenire su questo: il punto è questo. Il dato vero è che non c'è una politica, non c'è un'idea, che purtroppo manca da tempo; mancava anche negli anni precedenti. Da molti anni in questo Paese non c'è una politica per la casa; c'è una politica che interviene, tentando di calmierare

è affittabile; bisognerebbe rimetterli a posto, perché questi sì che diventerebbero un elemento di calmierazione, oltre che di risposta ai fabbisogni delle persone in carne ed ossa.

affrontare il problema della morosità incolpevole e immediatamente la questione dei mutui, ma, nel frattempo, costruire anche una proposta in grado di mettere sul mercato un certo numero di alloggi (almeno 300.000 per quanto riguarda l'edilizia economica popolare).

mi pare sia chiaro a tutti che la problematica della casa non riguardi soltanto le fasce deboli, ma tutte tutte le componenti della popolazione, anche e soprattutto strategiche, come i giovani, gli studenti e le famiglie giovani, che saranno l'ossatura del futuro della nostra società. Non posso che condividere quindi la visione del senatore Magni: torniamo sempre a parlare nello stesso modo, cioè a dire che questi sono problemi particolarmente complessi, in una stagione particolarmente complessa della nostra esistenza, che quindi necessitano di piani e di un'idea di un'idea per venirne fuori. Ora vorrei soltanto ricordare brevemente che siamo nettamente il Paese d'Europa con il maggior numero di alloggi in proprietà,

pensiamo di poter andare verso un Paese in cui tutti sono padroni della casa con i mutui che potrebbero improvvisamente scoppiare e mettere tutti in ginocchio? O pensiamo invece che forse sarebbe meglio avere un pochino meno proprietari di casa? Capisco che il dio mattone attiri, però, ragazzi, se poi non si è in grado di mantenerla, la casa, o di farci manutenzioni costose per le quali non si hanno i soldi, la conseguenza è un patrimonio edilizio scadente e non in grado di essere recuperato. Sono riflessioni che vanno fatte in maniera evidentemente abbinata, quelle sul patrimonio edilizio e quelle sull'edilizia abitativa possibilmente agevolata per chi ne ha bisogno: è chiaro che lo stimolo che questa mozione vuol dare al Governo è perché cerchi di impegnarsi a fare,

ringraziando i colleghi del Gruppo Partito democratico per aver sollevato il problema, perché oggi la mia collega, senatrice Paita, diceva che, se c'è un tema veramente fondamentale, che dovremmo risolvere e affrontare assolutamente, perché

così importanti, se la sanità è il numero uno, la casa è sicuramente il numero due, per la semplice ragione che rappresenta nella vita di ciascuno di noi parte integrante e fondamentale del proprio progetto di vita. Non esiste un progetto di vita, se non ci

per moltissime ragioni. Potremmo davvero guardare a questo fenomeno da mille punti di vista. Il collega senatore Spagnolli faceva giustamente una riflessione tra affitti e proprietà: il tema della penuria di case in affitto e anche di una certa mancanza di abitudine culturale all'affitto, perché noi italiani tendiamo a comprare, è anche probabilmente una delle ragioni per le quali i nostri ragazzi stanno in casa fino a trent'anni. È evidente che se non c'è la possibilità di affittare, finché non hai l'età per poter acquistare, starai a casa con mamma e papà. Questo comporta sicuramente un problema da molti punti di vista, su come l'assetto della nostra società si modella, rispetto ai modelli di vita, rispetto all'investimento sul lavoro, rispetto anche all'indipendenza dei nostri ragazzi. Di questioni legate alla casa ne abbiamo tantissime. Il collega Magni giustamente richiamava la nostra attenzione sul tema delle case popolari e dell'edilizia popolare, ma sappiamo - perché è la verità

manutenzioni. Nella città nella quale abito, Milano, ci sono esempi di case popolari e di edilizia popolare mantenuta in modo molto preciso preciso e ordinato, ma anche esempi nei quali l'edilizia popolare diventa una specie di luogo nel quale è difficile addentrarsi, dove anche la sicurezza delle persone è a rischio. Vogliamo parlare delle nostre città? Ho detto che vengo da Milano e un altro tema è quello della gentrificazione delle nostre città, il fatto che ormai diventa sempre più difficile abitare i luoghi, trovare commercio di prossimità e vivere quelle città. Ancora una volta torna il tema della sicurezza, perché nelle città e negli spazi abitati c'è maggiore sicurezza. Questa è un'altra questione enorme. I prezzi salgono moltissimo perché diventiamo (questo non è necessariamente un male) un luogo di investimento, anziché un luogo dove la casa è acquistata per viverla; la città diventa un luogo in cui la casa è un investimento finanziario, magari con gente che viene anche da fuori ad investire. Non è male attrarre investimenti dall'estero, però certamente diventa un problema. Vogliamo parlare di mutui? parlare di mutui? È chiaro che ci sono questioni enormi. Tantissimi nostri concittadini stanno vedendo le loro rate dei mutui esplodere, ma noi come legislatori abbiamo da un lato la necessità di venire incontro a queste persone, dall'altro anche la necessità di stabilire la regola che non è che quando si fa una scelta finanziaria sbagliata arriva il contribuente e ti salva dalle sue conseguenze. È chiaro che se io avessi preso

da un lato occorre supportare chi si trova in difficoltà, dall'altro però occorre stabilire che c'è una responsabilità nelle scelte fatte. Dico tutto questo per dire che alla fine ci asterremo, che lo strumento che è stato utilizzato sia quello sbagliato. Cioè, il tema della casa è un tema talmente grande che meriterebbe probabilmente una sessione dei nostri lavori e ho fatto soltanto qualche esempio. Il dialogo tra PD e Governo, che ha dovuto fare un lavoro di cesello, per

ci tiriamo fuori da questa dinamica, che non ci sembra quella corretta. Ringraziamo il PD per avere acceso un faro su questo tema e chiediamo al Governo e al resto delle forze politiche di aprire una sessione di riflessione autentica su una questione che ci riguarda tutti. Ci presenta delle premesse che partono dallo stato dei fatti, dimenticandosi di citare che i dati degli anni precedenti coincidono con gli anni di governo del centrosinistra. Ecco quindi che i 19 impegni della mozione, che corrispondono ad altrettanti interventi legislativi nell'ambito della casa, che ci propone il PD, praticamente sono un promemoria di quello che in tanti anni di governo la sinistra non è riuscita o non ha voluto o non ha voluto realizzare. La realtà è certamente più complessa, ma allo stesso tempo mostra il differente tipo di approccio che hanno il centrodestra e il centrosinistra sulla casa, anche se su alcuni punti concordiamo. Il punto di vista del centrodestra è certamente a favore della tutela della proprietà privata, quello di agevolare l'acquisto di una casa e di ridurre il peso della tassazione sia sulla proprietà che sugli affitti. In questo modo si rendono disponibili più immobili sul mercato e si ha un effetto positivo, anche sulla loro disponibilità numerica e sugli affitti che diventano così Il contrario in pratica di quello che voleva fare la sinistra, rivedendo gli estimi catastali con il conseguente aumento delle tasse che si ripercuote sul livello degli affitti. La possibilità di avere una casa di proprietà deve essere un diritto. Per questo stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti per agevolare l'accesso all'abitazione da parte di tutti, *in primis* sicuramente i giovani. Allo stesso tempo, pensiamo che le politiche abitative devono prevedere strumenti di edilizia popolare per chi non possa accedere alle case di proprietà; sicuramente un nuovo piano casa, ma per aiutare le case popolari bastano anche dei piccoli interventi. Vi sembra normale che le case popolari debbano pagare l'IMU come se fossero seconde case? Da tanti anni Federcasa ci chiede di mettere a posto

Il programma innovativo della qualità dell'abitare, che stiamo implementando e che verrà realizzato con i fondi del PNRR, pari a circa 2,8 miliardi, prevede la realizzazione di 10.000 unità abitative con 800.000 metri quadrati di spazi pubblici interessati. Sulla rigenerazione urbana, tra l'altro, a settembre inizierà l'esame in 8a Commissione della proposta di legge di Forza Italia, a prima firma del senatore Gasparri. La situazione post-Covid e la crisi energetica conseguente all'invasione dell'Ucraina ci ha costretto a investire risorse, decine di miliardi, per sostenere le famiglie in modo tale che potessero utilizzare servizi essenziali come il riscaldamento e la luce elettrica. Nonostante questo, nella manovra di bilancio sono stati prorogati molti incentivi per il mondo della casa, come l'ecobonus, il sismabonus, il *bonus* verde, il *bonus* barriere architettoniche e gli incentivi fiscali previsti per l'acquisto della prima casa per i giovani *under* Sono state introdotte anche delle novità. Ad esempio l'aumento del *bonus* mobili, la detrazione del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di case *green*, la rinegoziazione del mutuo passando da tasso variabile a tasso fisso e l'esenzione IMU per immobili occupati. In questi mesi di governo abbiamo anche chiuso l'enorme falla nei conti pubblici provocata dal MoVimento 5 Stelle e dal suo fallimentare 110 Per il futuro il Governo sta preparando un provvedimento per razionalizzare il sistema dei *bonus*, inserendo aiuti per le famiglie in difficoltà e per gli incapienti. Superata la crisi energetica, che ha assorbito, come dicevamo, risorse enormi, aumenteremo ulteriormente gli interventi nel settore casa. La maggioranza di centrodestra ha ben chiaro il percorso per valorizzare la casa e tutelare tutti gli attori del settore, dai proprietari agli inquilini, dalle imprese agli artigiani, dai lavoratori alle case popolari. Nell'azione di governo e nel lavoro parlamentare continueremo a seguire quanto contenuto nel nostro programma, quello che ci ha fatto vincere le elezioni, che vede la tutela della casa al centro della nostra azione politica. Per questi motivi, annuncio il voto contrario di Forza Italia, a malincuore, perché le proposte avanzate dal vice ministro Bignami erano sicuramente ragionevoli. la mozione a prima firma del senatore Mirabelli, che colgo l'occasione per salutare affettuosamente anche se non è presente in Aula *(Applausi)*, ci dice prima di tutto che il Governo è fermo sulle politiche abitative. Vice ministro Bignami, il ministro Salvini annuncia un piano casa ogni tre ore: lo ha detto a dicembre, lo ha ripetuto a gennaio, lo ha detto di nuovo a marzo, lo ha detto quindi a giugno e poi lo ha ripetuto di recente, annunciando un piano casa per il prossimo autunno. In ossequio alla prassi adottata da questo Esecutivo nelle ultime settimane, se non abbiamo le risposte e se siamo in difficoltà ci rimandiamo a settembre, come si fa con gli scolaretti. Ma quando si viene rimandati a settembre la prima cosa da fare è mettersi a studiare e non mi pare proprio che questa sia la strada da voi intrapresa. *(Applausi)*. Gli italiani vi hanno promosso una volta, sì, è vero, ma non si può pensare di passare all'anno successivo se ci si fa trovare costantemente impreparati su ogni cosa e qui invece siamo al paradosso che chi ha deciso di investire nella propria formazione, chi ha voglia di studiare deve combattere e fare continui e pesanti sacrifici per potersi permettere un'abitazione. I dati contenuti nelle premesse di questa mozione sono davvero allarmanti ed evidenziano la necessità di agire in fretta, senza tentennamenti. Come MoVimento 5 Stelle in questi anni abbiamo più volte richiamato l'attenzione sui bisogni e sulle necessità dei ceti meno abbienti, oggi più che mai costretti a combattere ogni giorno contro il caro mutui e il caro affitti. La nostra Costituzione, al contrario di quanto fanno quelle del Belgio, del Portogallo, della Spagna e della Svezia, non riconosce espressamente il diritto all'abitazione, anche se la Corte costituzionale fin dagli anni Ottanta lo ha qualificato come diritto sociale fondamentale. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono fondi per questo tema e per questo settore. Il Piano rappresenta un'occasione senza precedenti, ma deve essere percepito e usato come potentissimo strumento a disposizione del nostro Paese. Mai come in questo periodo storico abbiamo la possibilità di di ridurre le disparità e le disuguaglianze grazie al PNRR. Mentre qualcuno parla di autonomia differenziata per accentuare ulteriormente i divari preesistenti e magari crearne di nuovi, noi del MoVimento 5 Stelle ci concentriamo sull'esatto opposto e crediamo fortemente in una nuova concezione e visione delle politiche abitative. Tornando alla mozione che ci apprestiamo a votare, la richiesta di rifinanziamento del fondo affitti, cosa che qualcuno evidentemente ha dimenticato di fare. Positivi sono anche le proposte sulle rate dei mutui e gli interventi di rigenerazione urbana, così come indicato negli obiettivi previsti dalla missione 5 del PNRR. Condividiamo le richieste di potenziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, quelle finalizzate all'attento monitoraggio e sostegno all'utilizzo del superbonus 110 per cento, per il quale si chiede di valutare l'opportunità di una proroga dei termini per la realizzazione degli interventi.

formulata al Governo è quella di finanziare e realizzare un programma nazionale pluriennale di edilizia residenziale pubblica, ovvero un piano casa, a consumo di suolo zero. Il suolo è un bene primario non rinnovabile e su questo c'è bisogno di nuova consapevolezza davvero da parte di tutte Nella mozione n. 65 il senatore Mirabelli fa riferimento al potenziamento dell'offerta di edilizia residenziale universitaria pubblica. Ogni commento su questo punto è superfluo: sappiamo bene cosa è accaduto nelle ultime settimane. La vostra impreparazione è costata al Paese mezzo miliardo di euro: parlo della terza rata del PNRR. Dite che siete in grado di recuperare a settembre. Sì, come gli scolaretti. Andrà meglio?

Mi associo infatti alle osservazioni di chi poc'anzi riteneva opportune le modifiche che sono state proposte dal Governo, ma questo non cambia nella sostanza un atteggiamento di sensibilità che credo la Lega possa dimostrare di avere e di aver avuto, anche grazie a tanti suoi amministratori.

ti porta necessariamente a stare vicino ai problemi che ricordava la collega. La Lega conosce molto bene quei problemi per aver purtroppo ereditato la gestione di città e aver preso molti voti in quei quartieri popolari dai quali arrivano la stragrande maggioranza delle problematiche che poc'anzi i colleghi di sinistra stavano ricordando. Purtroppo, però, quei problemi non li possiamo risolvere con la bacchetta magica: sono questioni che vanno risolte col pragmatismo e con tante risorse. Questa è la verità. Da amministratori quali noi della Lega storicamente siamo,

delle istanze che provengono da tante aggregazioni e sodalizi che sui territori affrontano i problemi quotidiani dell'abitare. Da quell'incontro è emerso che ci sarà un tavolo *ad hoc* in cui si discuterà dell'emergenza abitativa e si parlerà di sfratti e anche del finanziamento (forse in legge di bilancio) della morosità incolpevole e probabilmente anche del monitoraggio sul piano della qualità dell'abitare.

quando si lavora a stretto contatto, come amministratori, con le proprie comunità. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il senso della mozione che abbiamo voluto presentare oggi, a proposito della quale ringrazio il senatore Mirabelli per il lavoro costante e continuo fatto in quest'Aula, ma anche fuori da quest'Aula su questo tema *(Applausi)*, è quello di promuovere una svolta sul tema del diritto alla casa, ma soprattutto di rimetterlo all'ordine del giorno. Una svolta e rimetterlo all'ordine del giorno. Si tratta di un tassello importante di quel *welfare* di cui oggi le opposizioni hanno voluto parlare, mettendo all'ordine del giorno la questione della sanità, del salario minimo, dei LEP, del significato dell'autonomia differenziata e adesso il tema della casa. Da un lato la pandemia di Covid e la crisi economica hanno peggiorato il quadro, aggravando l'emergenza abitativa; dall'altro sono cambiate le esigenze abitative, che necessitano di risposte diversificate a sostegno dei bisogni, ma anche dei progetti di vita. Si diceva prima che il punto è dove vogliamo andare, dove vuole andare questo Paese, guardando ai bisogni delle persone. Pensiamo solo - l'ha detto prima anche la senatrice Zambito - a come sia importante questo tema per una delle questioni che questo Governo a parole afferma di voler affrontare, cioè la denatalità; come sia importante per l'autonomia dei giovani e delle ragazze, per l'uscita da casa. Però bisogna fare i conti con i cambiamenti: come è cambiato l'abitare, ma anche come è cambiato il ruolo che la casa ha nei percorsi di vita delle persone. Quella della casa è una grande questione di interesse pubblico, questo abbiamo voluto dire. *(Applausi)*. Una grande questione di interesse pubblico nazionale, che non si può delegare a un gioco di domanda e offerta, né solo a politiche locali, perché ci sono buone pratiche di politiche locali, ma non possiamo lasciare soli gli enti locali, i Comuni, ad affrontare questo tema. Vorrei ricordare che nel 2016 noi mettemmo 490 milioni per recuperare 6.000 alloggi non utilizzati, a sostegno dei Comuni. *(Applausi)*. Non si parte da zero su questo punto, ma ci vuole un salto di qualità. Ce lo chiedono i cambiamenti ce lo chiede il modo nuovo di guardare alla casa, che non è solo la casa, ma è l'ambiente, gli spazi comuni, i servizi, il vivere urbano, il vivere delle persone. Per questo come Partito Democratico abbiamo parlato di un vero e proprio piano casa: 19 punti che ha illustrato la collega Zambito. Mi piace citare qui il senatore Mirabelli: quello della casa è un bisogno prioritario per ogni famiglia e purtroppo è diventato un problema per molti, per chi non è nelle condizioni di potersi permettere di sostenere un affitti e per chi è costretto, dovendo sostenere costi che aumentano, a destinarvi una parte sempre più importante e insostenibile del proprio reddito. reddito. Ma il problema è che la politica continua da anni a non mettere il tema tra le priorità e l'assenza di politiche pubbliche sulla casa fa sì che i problemi si aggravino. E si sono aggravati. A maggio la questione è esplosa grazie alle proteste delle tende degli universitari contro il caro affitti e per il diritto allo studio. Non mi pare che il Governo abbia assunto e recepito davvero fino in fondo quello che gli studenti hanno detto. *(Applausi)*. Non c'è infatti solo il tema della rata e dei fondi che abbiamo risparmiato adesso e rimesso nella quarta. Il punto è che c'è un problema di manutenzione delle residenze pubbliche, che negli anni si sono deteriorate.

La protesta esplode - me lo faccia dire, Presidente - perché ci sono già state delle scelte di questo Governo, visto che ormai governate da un anno. C'è già stato un bilancio fatto da voi e voi avete azzerato

"possiamo vedere", "valuteremo". Il segnale non può essere che non scegliamo il consumo zero di suolo. Queste politiche, infatti, vanno fatte non consumando più suolo pubblico *(Applausi)*, investendo nel nostro territorio e nel Parlamento che abbiamo. sapendo che, come ci dice il Parlamento europeo nella sua risoluzione, quello a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili è un diritto, una condizione preliminare per altri diritti fondamentali: questo volevamo dire oggi.

diritto alla casa non è una cosa che inventate voi in questa mozione, che tra l'altro apprezzo e di cui do atto al senatore Mirabelli. Pensate - per chi non lo sapesse - che già nel 1903 il deputato Luigi Luzzatti, con la legge del 31 maggio 1903, n. 251, istituiva una legge a favore delle case popolari. Sono passati centoventi

affrontare insieme un grosso problema che effettivamente mai era stato affrontato. Siamo infatti di fronte a una serie di problemi che sono cambiati nel tempo: è stato detto bene. Le esigenze sono cambiate, ci sono case che non sono più adeguate alle esigenze attuali sia per dimensioni, sia per consumi energetici, sia per inadeguatezza, che negli anni si sono sommati nelle abitazioni popolari: 837.000 abitazioni gestite da 74 tra enti pubblici e aziende territoriali. C'è un problema che nessuno ha citato se non

organizzazioni criminali per far sì che persone occupino ingiustamente abitazioni che spetterebbero a tante persone che da anni attendono che venga loro assegnata una casa popolare.

anni? Dobbiamo comunque porre fine - e questo sarà un nostro impegno - a quello che mi auguro venga quanto prima considerato un reato, cioè l'occupazione della casa pubblica *(Applausi)*, un reato i cui colpevoli vanno espulsi dalla casa che ingiustamente occupano per dare spazio a tante famiglie che attendono. attendono. Colleghi del PD - e faccio un accenno anche alla senatrice De Girolamo, che gentilmente in maniera simpatica ha voluto in qualche modo tacciarci scolaretti impreparati - senatrice, colleghi della sinistra, colleghi dell'opposizione, noi non siamo scolaretti, assolutamente impreparati, ma siamo responsabili. Non vogliamo percorrere quella politica che voi questa sera, purtroppo, state attuando, quella degli sbruffoncelli che vanno a raccontare le favole al vicino di banco o a chi sta fuori, ai cittadini. Noi abbiamo la responsabilità ben chiara - e il vice ministro Bignami lo ha detto di collaborare per arrivare a risolvere un problema attraverso un piano casa che quanto prima attueremo, attraverso i fondi del PNRR che andremo a stanziare a tal proposito, in un percorso che non è semplice, che per anni è stato trascurato e non è certo attraverso questo sistema, che voi stasera state dando dimostrazione di perseguire, con una politica populistica e demagogica, che risolveremo i problemi delle case popolari. Ci costringete perché rifiutate la collaborazione, a esprimere un voto contrario in attesa che il buonsenso prevalga su di voi.

quella sulla direttiva UE sull'efficientamento energetico degli edifici, quella sugli impatti della normativa europea in materia di transizione energetica e ultima, ma non ultima, quella sul riconoscimento dell'Holodomor come genocidio ai danni del popolo ucraino. Queste

Femminista, protagonista delle battaglie per i diritti delle donne in Italia e nel mondo, esperta di cooperazione internazionale: il mondo era il suo orizzonte e le donne di ogni luogo, storia e cultura erano le sue sorelle. Nata ad Arezzo, ha studiato a Firenze. È arrivata poi al femminismo romano nel *Collettivo* di via **Pompeo Magno** e da allora è sempre stata in prima linea fino al Gruppo del mercoledì e al Centro documentazione Bianca Pomeranzi è stata una femminista importante, esperta del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne, una delle donne che hanno animato la Conferenza di Pechino delle Nazioni Unite nel 1995,

Bianca Pomeranzi è riuscita a essere una protagonista del movimento femminista lesbico, attenta al dibattito pubblico, alle politiche istituzionali, alla dimensione internazionale e alla complessità culturale del mondo. Lo spiegò lei stessa il suo impegno nella cooperazione internazionale: il punto dirimente era la possibilità di trovare corrispondenze tra donne di mondi allora molto lontani. Per farlo occorreva impegnarsi e tradurre in realtà quello che l'immaginazione suggeriva. La realtà: iniziò così a frequentare le istituzioni internazionali, lavorò alla nascita della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari women (Cedaw) appunto fu la prima delle elette, la più votata; un grande successo per l'Italia e per lei. Per tante di noi, Bianca è stata una maestra, simpaticissima, con un grande senso dell'ironia, attenta alle giovani generazioni e anche ai destini della sinistra, animatrice del animatrice del Gruppo del mercoledì, a cui va il nostro abbraccio. Un grandissimo abbraccio va alla sua compagna, la scrittrice Maria Rosa Cutrufelli. Come ho già avuto modo di dire, Bianca è già nella storia delle donne del mondo intero.

perché per la seconda volta in meno di otto mesi è stata aggredita da una persona che voleva più attenzioni di quelle che le erano state concesse: sua mamma era lì controllata, ma ugualmente ha perso il senno e la volontà di fare qualcosa di buono. Vengono distrutti i pronto soccorso e viene aggredito il personale sanitario: in tutto questo, si chiede